Senatori, desidero rivolgere un commosso pensiero di vicinanza ai familiari, ai colleghi, agli amici dell'ex senatore Romano Misserville. Uomo di grande apertura intellettuale, avvocato brillante e apprezzato giurista, Romano Misserville è stato un politico appassionato, rispettoso delle istituzioni e sempre attento alle istanze dei cittadini; senatore per quattro legislature, dal 1987 al 2001; Vice Presidente del Senato nella XII legislatura; autorevole componente delle Commissioni affari costituzionali, affari esteri e agricoltura, oltre che della Commissione parlamentare antimafia e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Nel corso del suo lungo impegno parlamentare, Romano Misserville seppe sempre contraddistinguersi per competenze, rigore professionale e costante apertura al confronto costruttivo. Profondo il legame con i territori del Lazio, con la Provincia di Frosinone in particolare, che Romano Misserville ha messo al centro di molte iniziative da lui promosse per lo sviluppo economico e la tutela delle risorse ambientali. La sua progressiva transizione dalle forze politiche della destra italiana a quelle di centro non ha mai messo in discussione la coerenza delle idee e l'onestà intellettuale. Con Romano Misserville ci ha lasciato un politico di razza, un galantuomo di grande carisma e di profonda umanità; una figura sopra le righe lo conoscevo bene - irriverente talvolta, protagonista di gesti eclatanti, anche in quest'Aula, ma certamente animata sempre dalla volontà di non far mai mancare il proprio impegno e le proprie capacità per lavorare bene nell'interesse esclusivo dell'Italia e degli italiani. In ricordo del senatore Romano Misserville invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Signor Presidente, la scomparsa del senatore avvocato Romano Misserville - come lei ricordava Vice Presidente del Senato della XII legislatura, ha suscitato un unanime compianto e un sincero cordoglio, molto più vasto del mondo politico della nostra Provincia, proprio per la singolare personalità - lei lo ha conosciuto - del senatore defunto. Brillante avvocato, vero principe del foro, aveva fondato la sua professione su una conoscenza approfondita del diritto penale, radicata in una vastissima cultura umanistica di cui faceva sfoggio ammirevolmente nelle aule dei tribunali di tutta Italia. Ugualmente nell'attività politica seppe ben presto emergere non solo per le sue eccezionali qualità oratorie, ma anche per la sua capacità di saper attrarre il consenso di vaste aree dell'elettorato non strettamente riconducibili alla destra italiana. Rieletto più volte in Senato - come lei ricordava - per quattro legislature, seppe accortamente allacciare rapporti di stima e collaborazione con colleghi provenienti da vari orientamenti politici, raccogliendo simpatie e attenzione dai più disparati gruppi, con una visione ampia e moderna dell'attività parlamentare. Tutti ne conserviamo il ricordo di una figura davvero fuori dal comune: un politico attento alle esigenze del territorio, ma nello stesso tempo pronto a interpretare al meglio le istanze di una politica nazionale fondata sugli alti valori di rispetto delle istituzioni e vero amore per la patria. L'unanime commozione per la scomparsa del senatore Misserville, che in questa Aula aveva fatto risuonare la sua voce in memorabili e applauditissimi interventi, è la migliore espressione della sua generosa dedizione alla cosa pubblica,

due episodi su tutti: il primo quando fu eletto per la prima volta nel 1987. Il nostro era un feudo democristiano e soprattutto andreottiano: quell'elezione fu una soddisfazione incredibile per la destra ciociara. Il secondo mi viene in mente proprio perché

quella mascherina che tutti noi mal sopportiamo e dobbiamo portare per forza - per portare all'attenzione di tutti il problema della Valle del Sacco, l'inquinamento ambientale delle nostre terre.

mercoledì scorso all'età di ottantasei anni, presso l'ospedale di Frosinone - come ha ricordato l'amico e collega Ruspandini - è morto il senatore emerito Romano Misserville. Avvocato penalista dal 1959 e cassazionista dal 1978, Misserville è stato attivamente impegnato in politica nella destra ciociara, fondatore del movimento politico Destra di Popolo; è stato cofondatore e presidente della camera penale, sezione di Frosinone. Venne eletto Vice Presidente vicario del Senato, come ha ricordato il presidente Alberti Casellati; nel 2004 è stato insignito del riconoscimento della toga d'oro.

Era una persona elegante, aveva un umorismo raffinato e colto e chiunque lo ha conosciuto ha potuto apprezzare la dedizione totale per il lavoro al servizio della comunità, della sua comunità in particolare, e del Paese, nonché la sua straordinaria capacità di conciliare il ruolo di avvocato e l'impegno politico. Nella sua omelia, don Tommaso Antonetti ha detto di Misserville che era tanto rumoroso in vita quanto silenzioso nell'ultima ora. E poi ha riportato le parole del nipotino proprio pochi giorni fa, aveva pronunciato sul nonno: quanto mi piace il modo di vivere di mio nonno, sa vivere con allegria e leggerezza, è un uomo colto e molto simpatico; ama la vita e i cavalli;

rivolgo le mie più sentite condoglianze, nel ricordo di un uomo che è stato un protagonista nella storia politica, sociale e culturale in particolare del territorio di Frosinone *(Applausi)*.

Romano Misserville nel corso della sua intensa militanza politica, sempre caratterizzata da una grande franchezza di posizioni. Esordì in quest'Aula nel 1987 indossando una maschera antigas perché voleva denunciare, al suo esordio dell'attività parlamentare, l'inquinamento che colpiva alcune zone del frusinate alle quali è sempre stato legato: lì ha vissuto e lì ha svolto con con grande valenza (e non sono nel frusinate) la sua attività forense, che ha sempre condotto con grande qualità e, anche fino ad anni recenti, affrontando vicende complesse, eclatanti, che hanno anche dominato le cronache

di vicende polemiche o controverse. Partecipò, sempre con uno spirito di grande autonomia, alla trasformazione della destra, alla nascita di Alleanza Nazionale, coniugando un impegno nel Parlamento e sui grandi temi della politica a una forte

perché era l'unico luogo dove non si trovavano asini. Era anche un uomo di battute sferzanti e di grande dialettica. Fu colpito anni fa dalla scomparsa prematura della figlia Fiammetta, che certamente ha segnato la sua vita, perché per un padre è sempre motivo innaturale

di alta professionalità, che però viveva la vita quotidiana del territorio, dei cittadini, dell'ascolto, coniugando professione, politica, territorio e Parlamento. Con questo spirito il Gruppo Forza Italia si associa alle sue espressioni, Presidente, ed esprime la propria vicinanza alla famiglia del senatore Misserville e a tutta la comunità territoriale che lo ha conosciuto e apprezzato

politico che è diventato! Egli incantava quando parlava e il suo modo di fare era legato a un linguaggio ricco di cultura, visto che sapeva sia di arte che di letteratura. Noi eravamo veramente

Egli aveva gesti convinti ed era un uomo libero, tant'è che preferì rinunciare all'incarico di Sottosegretario nel secondo Governo D'Alema, di cui aveva notevole stima, perché non volle togliere un quadro di Mussolini dalla sua stanza. Egli era molto convinto, ma mai fanatico, sempre pacato ed educato. Aveva una memoria straordinaria: conosceva

il suo cane, un pastore belga che lo sta ancora aspettando. Ceccano e Frosinone perdono «il senatore» e anche l'Italia perde un pezzo di storia. Rendiamo onore alla tua memoria, Romano, e che la terra ti sia lieve. *(Applausi)*.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

ci troviamo ancora una volta a dover contestare la costituzionalità dei provvedimenti che tendono a restringere, tramite il i diritti costituzionalmente garantiti, in particolare quelli legati alla libertà individuale e personale di ciascuno dei cittadini italiani. Noi continuiamo a essere fermamente contrari all'idea che, attraverso lo strumento del decreto-legge, si possa ipotizzare di limitare limitare diritti costituzionalmente garantiti. In particolare, il decreto-legge, il n. 2 del 2021, di fatto proroga fino al 30 aprile di quest'anno il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei due decreti emessi nella stessa identica direzione nel corso del 2020, e cioè il decreto-legge n. 19, che noi abbiamo fermamente contestato, e il decreto-legge n. 33, che ha parzialmente ridotto i i difetti costituzionali contenuti nel primo, appunto il n. 19. Continuiamo a essere fermamente contrari all'idea che i cittadini italiani possano veder ridotta la possibilità di muoversi all'interno della propria città, della propria Provincia o della propria Regione esclusivamente con un provvedimento del Governo. Noi riteniamo che questo non sia possibile. Tra l'altro, aggiungo che il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, 21 maggio 2020, ebbe a dichiarare, proprio in quest'Aula, che non ci possiamo permettere - recito le sue parole di protrarre l'efficacia di misure limitative per un tempo indefinito. Un ordinamento liberale e democratico non può, infatti, tollerare una compressione dei diritti fondamentali, se non nella misura strettamente necessaria a difendere i beni primari della vita e della salute dei cittadini, in dipendenza di una minaccia grave e attuale. La permanenza di misure così severe sul piano delle limitazioni dei diritti fondamentali, oltre il tempo necessario a invertire la curva del contagio,

avere una misura temporale senza limiti chiari e definiti non è ipotizzabile (la nostra Costituzione non lo consente). Se si parla di decretazione d'urgenza, si fa esclusivo riferimento a provvedimenti che devono avere una limitata azione nel tempo e una limitata efficacia nel tempo. Voi capite bene, però, che tutto questo non sta accadendo. Aggiungo nel merito - come anche altri colleghi, e non solo del mio movimento politico, affermato in questi giorni - che i provvedimenti di limitazione della libertà individuale - mi riferisco, per esempio, al cosiddetto decreto Natale - non hanno prodotto alcun giovamento in termini di contagio. Abbiamo potuto constatare che l'aver rinchiuso le persone nelle proprie abitazioni non ha impedito che il contagio continuasse a correre. Quindi, anche nel merito, non ha senso non ha senso persistere con limitazioni di siffatta natura. Capisco ed è necessario che si vada avanti con un progetto nazionale di vaccinazione, con un piano che, nel più breve tempo possibile, possa permettere di vaccinare tutti, ma così non si può andare avanti. È il sistema che è sbagliato. Mi sono poi un po' stancato di riferire ogni volta che in questa Camera dobbiamo difendere le prerogative del Parlamento. *(Applausi)*. Non possiamo continuare a permetterci di violare regolarmente i principi costituzionalmente garantiti. Non mi stancherò mai di ricordarlo, e faccio bene a farlo qui. Concludo, citando un aspetto che oggi non solo è attuale ma cambia anche completamente le carte in tavola. Ieri è accaduto un fatto non secondario, caro collega Alfredo Messina. Ieri - come lei sa - abbiamo assistito a un voto che non dà

ha un senso se esistono maggioranze assolute nelle due Camere. *(Applausi)*. Siccome da ieri questo elemento non esiste più - in questa Camera la maggioranza è solo relativa

Signor Presidente, il Senato è chiamato oggi a convertire l'ultimo decreto-legge emanato dal Governo per far fronte alla crisi sanitaria in atto. Il provvedimento si inscrive in una complessa sequenza di atti normativi, spesso di difficile comprensione da parte dei cittadini, data la loro sovrapposizione e la continua contraddizione tra i diversi testi pensati per affrontare l'epidemia. Il decreto-legge è stato emanato in simultanea rispetto all'ennesimo DPCM, una fonte giuridica perlopiù sconosciuta fino a pochi mesi fa e diventata oggi la pietra angolare della normazione nazionale; una forma subordinata, spesso assurta impropriamente al rango primario, per la disciplina di una materia così delicata quale è la libertà personale; una modalità di produzione normativa su cui, come Italia Viva, abbiamo già più volte espresso le nostre perplessità; perplessità che possiamo riassumere nel fatto che il Parlamento è stato chiamato, il più delle volte, a convertire in legge un decreto-legge che altro non faceva che riproporre a sua volta una fonte subordinata quale è il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

attraverso una fonte subordinata rispetto a ciò che la Costituzione diversamente prescrive, come materia sulla quale la riserva parlamentare legislativa dovrebbe invece essere assoluta. Inoltre, una siffatta produzione normativa, confusionaria sul piano della gerarchia delle fonti, comporta anche conseguenze problematiche sul piano del lavoro parlamentare, relegando il Parlamento a un ruolo ancillare rispetto a decisioni assunte in altre sedi. Con il decreto-legge n. 19 del 2020 è stata - ad esempio - prevista la possibilità, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di gestire la complessa fase dell'emergenza sanitaria ammettendo di fatto - tramite una fonte primaria - che il Capo dell'Esecutivo possa intervenire attraverso una fonte secondaria, arrivando a stabilire limitazioni della libertà personale, per la cui disciplina vige una riserva di legge assoluta. Sulla base di tale postulato della gerarchia delle fonti - lo si ricorda - una fonte subordinata non può incidere su limitazioni della libertà personale. Al contrario, già da tempo, nell'attuale fase emergenziale, si assiste ad interventi normativi su questa materia, attraverso decreti del Presidente del Consiglio, che di certo non sono ascrivibili al livello di fonte primaria. Su questo tema il Parlamento, come abbiamo già osservato in Commissione affari costituzionali, dovrebbe compiere una riflessione approfondita, magari per ipotizzare una riforma del sistema, perché si pone una questione di peso: come può il Parlamento, in sede emendativa, modificare una fonte subordinata quale è quella contenuta in un DPCM, quando la fonte non è pedissequamente trascritta nel decreto-legge? In più occasioni, emendamenti che cercavano di modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati dichiarati inammissibili, perché modificativi di una fonte subordinata alla legge.

sessanta giorni, il Parlamento è chiamato a convertire. Poi però le parti estranee al decreto-legge, ma contenute nel DPCM, rimangono precluse dall'esame, perché non allineate sul piano della gerarchia delle fonti. In sostanza si tratta di un doppio *vulnus* al ruolo del Parlamento, sempre più spettatore rispetto alla gestione emergenziale. Per questo motivo, il Gruppo Italia Viva non può che sollevare forti perplessità in merito a questa modalità di produzione normativa. Chiediamo dunque che ci sia una riforma del sistema, che veda un ruolo più centrale del Parlamento nella gestione dell'emergenza e annuncio quindi un voto di astensione, a nome del Gruppo. *(Applausi)*.

Sulla proroga dello stato di emergenza, infatti, il decreto-legge in conversione si limita, correttamente, ad adeguare il quadro delle fonti primarie, che già disciplinano le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, alle specifiche esigenze che hanno condotto a tale proroga.

25 marzo 2020, n. 19, secondo il quale: «il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare (...), al fine di tener conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati».

la proroga dello stato di emergenza stabilisce il termine del 30 aprile, visto l'andamento preoccupante dell'emergenza epidemiologica da Covid e nel rispetto di quanto previsto dal codice della Protezione civile;

Non si ravvisa davvero alcuna ragione per definire atti normativi illegittimi i provvedimenti adottati fino a questo momento nell'assoluto rispetto del ruolo del Parlamento. In effetti, il ministro Speranza è venuto più e più volte a raccontarci qual è la situazione epidemiologica e quali provvedimenti avrebbero dovuto prendere, ovviamente sempre in sintonia piena con quello che dice la scienza. cambiamenti sono stati fatti, certo che sì, ma anche perché l'evoluzione epidemiologica ha influito tantissimo in questo periodo; nessuno sapeva come sarebbero andate le cose e bisogna ovviamente aggiustare il tiro ogni volta che ci troviamo di fronte a un'emergenza. Non si ravvisa davvero questo fatto. Quanto è previsto dalla Costituzione e dalle leggi viene rispettato in assoluta coerenza con il sistema costituzionale delle fonti e le logiche di equilibrio fra poteri che ad esso sono sottese. Tra l'altro, colleghi, vi ricordo che non tutti i nostri cittadini cittadini si lamentano. Ho parlato con tante persone che mi hanno detto che se dobbiamo fare un altro sforzo, lo facciamo proprio perché vogliamo essere più liberi dopo, senza il virus. Nessuno ha mai parlato di lesione del diritto alla propria libertà; i cittadini non vedono l'ora di essere liberi dal virus: questa è la vera

quante situazioni contrastanti abbiamo assistito, addirittura persone che siedono nelle istituzioni che vanno contro la legge: non si devono più vedere queste cose, perché i cittadini davvero si confondono. Dobbiamo essere anche su questo molto tesi per far capire che cosa si sta facendo. facendo. Complessivamente dobbiamo attenuare il rischio di un'epidemia non controllata e l'aggravarsi della pressione sulle strutture sanitarie. Vi ricordo che ancora adesso, purtroppo,

del virus. Stiamo facendo quello che è necessario fare per i nostri cittadini e credo che, per un'ultima volta, lo dobbiamo fare con questo DPCM. Siamo sicuri che riusciremo ad uscire perfettamente

chiarissimo, anche nell'esposizione degli interventi,

in un momento complicato della vita del Paese, non soltanto per la drammaticità, ma anche per il fatto che non è mai accaduto, nella storia repubblicana e credo nella storia di tutti i Parlamenti di costituzione democratica, di trovarsi di fronte a un evento così drammatico come la pandemia.

nell'affrontare soprattutto problemi di ordine di sicurezza nazionale. E questo è un problema di emergenza e di sicurezza nazionale. un equilibrio complesso dal punto di vista istituzionale che riguarda il rapporto con le Regioni e che ha scandito - negativamente e positivamente, a seconda dei momenti - tutte le fasi di questo lungo anno.

circa il fatto che, addirittura, si debba arrivare a una distribuzione dei vaccini in base al PIL delle Regioni (per comprendere a che punto siamo arrivati, anche di distanza nelle valutazioni). Si tratta di affermazioni molto gravi rispetto ai principi costituzionali e ai diritti dei cittadini, che sono

puramente ideologica. Per tutti questi motivi, respingiamo la questione pregiudiziale e la riteniamo assolutamente e certamente infondata.

signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 proroga al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza, confermando dal 16 gennaio al 15 febbraio il divieto di spostamento tra regioni e province; estende fino al 30 aprile 2021 la possibilità del Presidente del Consiglio di procedere con DPCM e si delega il Ministro della salute ad individuare, con una serie di parametri, alcune zone bianche in cui le restrizioni possono essere allentate; e, ancora, si prevede l'istituzione di una piattaforma informatizzata che possa servire a regolare il piano di vaccinazione. Siamo di fronte all'ennesimo decreto-legge, con l'utilizzo sproporzionato della decretazione di urgenza, che dimentica che nella nostra Costituzione non è contemplato un diritto speciale per lo stato di emergenza, come si evince in altre Costituzioni (quella (quella francese, quella spagnola o quella ungherese). In più, mi viene in mente l'informativa del signor Presidente del Consiglio del 21 maggio 2020, che voglio leggere - mi perdonerete - perché da essa partiamo per le nostre considerazioni. In quella circostanza il Presidente del Consiglio disse: «Non ci possiamo permettere di protrarre l'efficacia di misure limitative per un tempo indefinito. Un ordinamento liberale e democratico non può infatti tollerare una compressione dei diritti fondamentali, se non nella misura strettamente necessaria a difendere i beni primari della vita e della salute dei cittadini, in dipendenza di una minaccia grave e attuale. La permanenza di misure così severe sul piano delle limitazioni dei diritti fondamentali oltre il tempo necessario ad invertire la curva del contagio sarebbe dunque irragionevole e incompatibile con i principi della Costituzione». Benvenuto tra di noi, signor Presidente del Consiglio: è quello che noi sosteniamo. Nel momento in cui vengono contemperati illimitati diritti costituzionali fondamentali, non si può ricorrere in maniera indiscriminata a provvedimenti amministrativi come i decreti del Presidente del Consiglio. Ormai non siamo più di fronte a un'emergenza. Voglio ricordare che questa pandemia nasce nel gennaio 2020; è passato un anno non credo che il Governo abbia dimostrato di avere le idee chiare nel momento in cui avrebbe dovuto adottare non soltanto misure di prevenzione, ma anche misure di sostegno all'economia. C'è un grosso problema che viene dimenticato. Ci auguriamo tutti che il piano delle vaccinazioni parta come si deve, che ci siano forniture regolari, che ci siano anche altri vaccini omologati che possano allargare la platea dei prodotti da utilizzare. Ma, quando questa pandemia sarà stata sconfitta, non avremo terminato i nostri problemi, perché ci troveremo di fronte a una gravissima crisi economica, che questo Governo ha contribuito creare. È troppo semplice dire che, siccome c'è una pandemia e siccome non si allenta la curva del contagio, dobbiamo chiudere tutto. È troppo semplice; stanno nascendo proteste di attività produttive, che noi capiamo e che non condividiamo, perché siamo per il rispetto della legge. Signori miei, come si fa a spiegare a un ristoratore, che magari a febbraio, marzo o aprile dell'anno scorso, aderendo alle indicazioni di questo Governo, ha investito risorse importanti per rendere i propri locali adeguati alla pandemia, come si fa a spiegare a questi signori che negli alberghi si può consumare, che nelle mense si può consumare, ma nei ristoranti no, perché devono rimanere chiusi? Come fate a spiegarlo a queste persone disperate? E come fate a spiegare alle attività produttive, ai negozi, ai commercianti che devono rimanere chiusi, che devono decidere se morire di Covid o morire di fame? Non è questo quello che un Governo e una maggioranza seria dovrebbero attuare. I ristori, per quelli che li hanno avuti, hanno rappresentato sì e no il 7-8 per cento delle perdite, cosa ben diversa dal 70-75 per cento che altri Paesi, come la Germania, hanno messo a disposizione delle loro categorie produttive. Noi stiamo creando i presupposti di un Paese di poveri e di disperati, di una rivoluzione sociale. Di questo voi siete responsabili e non ci sembra che ci siano elementi di resipiscenza nella vostra attività legislativa. State bypassando le prerogative del Parlamento; facendo in modo di superare il dibattito e il confronto. Eppure dai banchi dell'opposizione, per bocca anche di autorevolissimi esponenti e *leader* dei partiti di opposizione, non una volta ma più volte

che la politica debba dare esempio di compattezza. Ci saranno momenti per le contrapposizioni, ci saranno momenti per le proprie diversità; oggi il Paese ha bisogno di unità e voi fate una crisi - vergogna! *(Applausi)* - in un momento così delicato, nel quale c'è gente che non riesce a portare a tavola qualcosa da mangiare per i propri figli e per la propria famiglia e non capisce perché, di punto in bianco, quello che andava bene ieri non va più bene oggi. Io credo che ci sia un limite che non possa essere superato e che anche voi conosciate: create i presupposti per una maggioranza coesa di Governo e assumetevi sino in fondo le vostre responsabilità oppure, diversamente, è inutile tirare a campare creando i presupposti per una situazione ancora più difficile da risolvere. che questa situazione l'abbiate creata voi e che voi dobbiate assumervene la responsabilità fino in fondo. Se non ne siete capaci, assumete le conseguenziali determinazioni, prima che sia troppo tardi. *(Applausi)*. La storia ci ha insegnato che le rivoluzioni non si fanno per questioni politiche, per contrapposizioni personali o per desiderio di *premiership*; si fanno per fame e l'Italia ormai è arrivata a queste condizioni. Assumetevi le vostre responsabilità. Per questo noi voteremo a favore della pregiudiziale di costituzionalità.

non perché non siamo convinti che siamo in una situazione di pandemia che debba essere affrontata attraverso alcune restrizioni per cercare di contrastare il contagio,

io penso che dopo un anno più che essere in emergenza uno Stato serio avrebbe dovuto almeno organizzarsi per affrontare la pandemia, contrastare e cercare di contenere il contagio. Ciò non è avvenuto

si cercano di attuare per migliorare la situazione sia sotto l'aspetto sanitario che sotto l'aspetto economico. Ripeto che non diciamo che le restrizioni

si tenessero aperti quelli che hanno più spazio e che possono rispettare maggiormente le distanze, quelli che sono obbligati a chiudere perché piccoli potrebbero ricevere indubbiamente maggiori ristori di quelli che normalmente vengono dati. Sono tante le valutazioni che si possono fare e invece voi andate avanti per la vostra strada. Chiudo riferendomi all'appello che ha fatto la collega, che ha detto che noi non capiamo nulla e che dobbiamo fare uno sforzo per essere liberi dopo. Questo è un ragionamento intelligente: facciamo un sacrificio oggi per essere liberi domani; però, a novembre ci dite che chiudiamo per

Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, è con un certo imbarazzo che intervengo oggi in quest'Aula e mi piacerebbe che lo percepisse anche chi parla disturbando il mio intervento. Sono in imbarazzo perché gli eventi di questi ultimi giorni ci hanno messo di fronte a un quadro completamente nuovo e ci obbligano, gioco forza, a distrarre il nostro sguardo e le nostre energie dall'unico vero fatto importante che dovrebbe impegnare tutte le nostre forze, maggioranza e opposizione, cioè il contrasto alla diffusione del virus e alla crisi economica che stiamo vivendo.

Questa sola considerazione dovrebbe essere sufficiente per ridimensionare quanto accaduto in questi giorni, eppure ci siamo trovati spesso, costretti dagli eventi, a parlare di ben altro. I rappresentanti dell'opposizione, anche oggi con questa pregiudiziale cercano di spiegarci in tutti i modi i motivi del loro dissenso. Al di là di tutti gli artifici retorici e di tutti i bizantinismi della politica italiana, di cui francamente mi dichiaro orgogliosamente inesperto, noi non stiamo affrontando uno scontro fra ideologie. Noi siamo qui per affrontare le conseguenze di una crisi sanitaria ed economica che dovrà ancora palesare tutti i propri effetti deleteri per molti anni ancora, con una coda che temo sarà molto lunga. Nel momento in cui bisogna caricarsi sulle spalle tutto il peso della gravità della situazione, la decisione di dividersi in seno alla maggioranza, come ieri avete visto tutti, a causa della crisi scatenata da Italia Viva, o di dividersi fra maggioranza ed opposizione non fa che indebolire l'azione di questo Governo a svantaggio dei cittadini, i nostri datori di lavoro,

non solo a parole. Va bene la critica, ma partecipate alle nostre scelte: i nostri figli, i vostri figli ve ne saranno grati. Del resto, gli eventi e la necessità

per loro, per la Lega come per il PD, vale per tutti, non solo in un senso. Eppure, il senso di responsabilità ci ha portati a superare le nostre divisioni e i nostri pregiudizi, pagando anche un prezzo importante all'interno della nostra formazione politica, alleandoci prima con la Lega e poi con le forze di sinistra. Dopo defezioni e scissioni, però, siamo ancora qui, noi, a guidare questo Paese, nell'ora più buia della sua storia recente. Perché lo abbiamo fatto? Perché lo stiamo facendo? Questa scelta ha dato risultati importanti? Certamente sì, ma non per il MoVimento 5 Stelle, non per il PD, non per LeU,

e avere ottenuto questo è un risultato importantissimo, aver ottenuto così tanto nella ripartizione del *recovery fund* è un risultato epocale; l'emissione di un prestito con l'emissione di un prestito con titoli di debito comune garantito dall'Unione si avvicina finalmente all'idea di un debito condiviso. Neanche due anni fa, cari colleghi, lottavamo per uno scostamento dello 0,4 per cento adesso invece siamo chiamati a portare a casa il *recovery plan*, che è il più grande investimento di risorse economiche del nostro Paese dalla Seconda guerra mondiale, un vero e proprio piano Marshall. Questo ulteriore provvedimento emergenziale, necessario per fronteggiare l'emergenza sanitaria, non ha bisogno adesso dell'utilizzo strumentale che fate delle pregiudiziali, bensì di una sana e robusta discussione fra maggioranza e opposizione, per migliorare

come mezzi eccezionali in un momento eccezionale, ma sempre nell'alveo della Carta. Prorogando lo stato di emergenza, dotiamo il Governo di tutti gli strumenti necessari per agire con tempestività ed efficacia. A chi ci accusava di essere contro l'Europa fino a ieri, noi abbiamo dimostrato che eravamo contro quell'Europa, l'Europa della rigidità contabile, dell'*austerity*, l'Europa che considerava i sussidi come uno spreco di denaro pubblico e che invece adesso ricorrere al sostegno pubblico all'economia, come sapete bene, e ai cittadini che sono anche i vostri cittadini, non solo i nostri, tramite i ristori in tutta Europa. Abbiamo dimostrato che un diverso rapporto con l'Unione è possibile, un rapporto sì conflittuale, ma sincero e responsabile, nell'esclusivo interesse di tutti i Paesi membri, nell'interesse di quell'Europa dei popoli che tanto sta a cuore a tutti noi, contro le politiche di *austerity* imperanti fino a pochi anni fa. Alla lunga, cari colleghi, questo impegno è stato riconosciuto e ha dato i suoi frutti grazie all'instancabile lavoro del presidente Conte, di tutto il Governo e del ministro Amendola in particolare. Tutto ciò non può andare perso adesso. Ora più che mai il Paese necessita di una guida solida, di una concordia inscalfibile tra le forze di Governo e lo sguardo vigile e però collaborativo dell'opposizione, perché da questa concordia, oggi più che mai, dipende il destino di tutta l'Italia. Abbiamo bisogno della forza per prendere altre scelte importanti e difficili e per sostenere quelle già prese. qui deriva la necessità di avere l'aiuto di tutti gli uomini e le donne di buona volontà di questa Assemblea, cui ieri si è richiamato anche il presidente Conte. In caso contrario, il prezzo da pagare potrebbe essere troppo alto e le conseguenze politiche e sociali imprevedibili. Il popolo italiano si è dimostrato paziente nel rispettare le severe norme che la pandemia ha imposto e le varie restrizioni sulla libertà personale, ma potrebbe sopportare una crisi di governo allo stesso tempo? Abbiamo appena visto che cosa è accaduto in una grande democrazia come gli Stati Uniti quando si è presentata solo la parvenza di un potere non legittimato. La debolezza della politica in questo momento fornirebbe in Italia linfa vitale a pulsioni antidemocratiche che, seppur striscianti nella nostra società, vediamo che sempre sopravvivono, se siamo però capaci di guardare oltre i vetri delle finestre di questi palazzi.

aggiungo anche coerenza nel presentarci al Paese con idee concretizzabili e risultati tangibili nell'esclusivo interesse dei cittadini. Scuola, sanità, lavoro e impresa non aspettano altro. Come ci si può dividere su questi temi? penso e non lo condivido. Il voto dell'Assemblea oggi, come quello di ieri ma anche come quelli futuri, metterà ciascuno di voi di fronte alle proprie responsabilità, davanti al Paese e davanti alla storia. Il prolungamento dello stato di emergenza e l'adozione di tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione dell'epidemia nasce da dati di fatto relativi all'evolversi della pandemia e all'incremento preoccupante dei casi positivi e dei decessi. Mai come adesso politica e scienza sono andate così bene insieme. Anche il voto che oggi pomeriggio ci apprestiamo a dare allo scostamento di bilancio chiamerà tutti noi, nessuno escluso, maggioranza e minoranza, a compiere delle scelte oltre la partitocrazia, oltre le proprie convinzioni e oltre le logiche dell'appartenenza a questa o a quell'area politica. Scelte operate nell'esclusivo interesse dei cittadini in questa greve ora. In caso contrario, veramente volete assumervi la responsabilità - direi la colpa davanti alla storia del Paese di continuare ad alimentare crisi agli occhi dei cittadini? Di fronte a tutto questo, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad una scelta di responsabilità.

L'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi e dei decessi ci impongono di frenare la contagiosità e lo sviluppo di nuovi focolai. Stiamo vivendo in un momento storico eccezionale. Stiamo cercando di governare le sorti con gli strumenti di cui disponiamo; la legge e la scienza; non abbiamo di meglio. In situazioni eccezionali anche le risposte devono essere pronte, chiare e improntate a fermezza decisionale e precisione. Proprio grazie alla prontezza con cui il Governo ha dichiarato il 31 gennaio 2020, come ricordava il collega, lo stato di emergenza si sono potuti mettere in atto tutti i provvedimenti necessari a contenere la curva dei contagi. Il Governo, nel raggiungere questo obiettivo, non ha mai esautorato il Parlamento che, al contrario, ha continuato sempre a svolgere le proprie funzioni. Stiamo discutendo un decreto-legge... AUDDINO *(M5S)*. Stiamo discutendo un decreto-legge che vedrà il giusto coinvolgimento del Parlamento, ricordando che siamo davanti a una situazione che richiede provvedimenti di assoluta necessità e urgenza.

Senatori, desidero invitare l'Assemblea a stringersi in un momento di solenne raccoglimento in ricordo del senatore Emanuele Macaluso. Nato a Caltanissetta il 21 marzo 1924, figlio di un operaio delle ferrovie e di una casalinga, Emanuele Macaluso si diplomò perito minerario, perché quella era la scuola che avevano frequentato i suoi fratelli e quelli erano gli unici libri disponibili in famiglia. È proprio negli anni dell'adolescenza che maturarono in lui la consapevolezza delle enormi difficoltà in cui versava la sua terra e la volontà di rimboccarsi le maniche, per aiutare Comunista Italiano, di cui divenne presto dirigente e figura chiave, in un'epoca complessa, di fragili equilibri economici e di profondi conflitti sociali. Parlamentare per ben sette legislature, dal 1963 al 1992, di cui quattro vissute tra i banchi del Senato, Emanuele Macaluso fu sempre un politico concreto e dialogante, caratterizzato anche da una grande libertà di pensiero e da una visione moderna e riformatrice dell'impegno politico.

Persino durante questi drammatici mesi di pandemia, Emanuele Macaluso non ha mai smesso di interessarsi alle vicende politiche e sociali italiane, di analizzarle e commentarle con incredibile lucidità. Con Emanuele Macaluso ci lascia un autentico protagonista di due secoli di storia nazionale, una delle più incisive coscienze critiche nella costruzione della nostra democrazia e nel consolidamento dei suoi valori. In ricordo del senatore Emanuele Macaluso, invito l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio.

Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere un omaggio molto sentito, affettuoso e deferente alla memoria di Emanuele Macaluso, una grandissima personalità di questi anni, della fine del Novecento e delle contrapposizioni ideologiche di quel secolo, e un attento osservatore della politica di oggi. Anche dall'alto di un'età veneranda, ha sempre dato giudizi particolarmente acuti, intelligenti e anticonformisti. Le sue odierne parole, signor Presidente del Senato, sono state la testimonianza migliore di quello che tutti noi pensiamo di Emanuele Macaluso. Mi consenta di aggiungere

di scontri, anche duri, ma su principi e valori ritenuti indisponibili. Emanuele Macaluso è stato questo e il fatto che al termine della sua vita,

chi vorrebbe commemorare Emanuele Macaluso è stato il suo grande amico, il suo compagno di mille battaglie politiche nel PCI e

ha lavorato con Togliatti, con Berlinguer e poi con Occhetto nel senso di una direzione riformista per il Partito Comunista Italiano. Ha lavorato in modo anticonformista negli ultimi anni per dare senso alla direzione di marcia di una sinistra che, dopo la caduta del Muro di Berlino, stentava a trovare la via giusta, ma soprattutto si è sempre speso a favore dei diritti di tutti, anche dei suoi avversari politici. Consentitemi, proprio a tal proposito, di terminare leggendo quello che Emanuele Macaluso scriveva,

Macaluso scriveva: «Quello ad Andreotti e all'andreottismo doveva essere un processo fatto dalla politica, capace di avviare una seria riflessione sui fenomeni che hanno distorto e a volte inquinato la Prima Repubblica. Invece si è celebrato un lungo processo penale che ha trascinato cinquant'anni di storia politica nel chiuso di caserme e procure. Con la conseguenza che, alla fine della giostra, il sipario della prescrizione è calato non solo su Andreotti ma su tutta la Democrazia cristiana, da De Gasperi a Scelba, da Fanfani a Moro fino a Rumor. Un'ingiustizia.». Emanuele Macaluso, con i suoi ottantanove anni, non si dava pace di questo e si sentiva in dovere morale di riportare sul piano della politica il giudizio che lo contrapponeva ai suoi avversari di prima, cioè alla Democrazia Cristiana, di cui era stato avversario, ma di cui ha sempre rifiutato ogni idea di criminalizzazione. Questo era lo scontro, colleghi (lo dico soprattutto ai più giovani), delle personalità di trenta o quarant'anni fa, che mai avrebbero pensato a scorciatoie di tipo giudiziario o a fatti di slealtà per contrapporsi gli uni agli altri in un dibattito che era invece animato da una grandissima passione civile. Per me Macaluso è stato un esempio, per me che mai ho militato nella sua parte politica, ma mi sento in questo senso di rivolgergli un ringraziamento, perché è stato veramente una personalità da cui soprattutto i più giovani, che si avviano alla politica, devono

Con la morte di Emanuele Macaluso perdiamo un pezzo di storia riformista della sinistra italiana; perdiamo, come è stato già detto, uno spirito anticonformista, un migliorista. Perdiamo una persona che ha dato veramente tutta la sua vita alla politica, prima nel sindacato e nel giornalismo, poi come dirigente del Partito Comunista Italiano;

all'interno delle nostre case, separati dagli altri e costretti a combattere la paura restando soli. Questa cancellazione della vita sociale influirà su ognuno di noi, Come giustamente ha detto in questa recente intervista, sappiamo quanto stiamo soffrendo per questa situazione che ci toglie ogni vita relazionale, la vita sociale cui siamo abituati; ma quella solitudine e quel silenzio di cui Macaluso parlava nelle ultime interviste erano il contrario della sua vita politica, quella di una grande personalità che ha segnato la storia della politica e della sinistra italiana, una coscienza laica e critica. La sua vita e la sua cultura politica hanno accompagnato periodi difficilissimi della storia italiana, quando era difficile essere un migliorista, insieme al suo grande amico Giorgio Napolitano. Macaluso era un uomo scomodo, come è stato prima ricordato, ma era sempre attento e protettivo verso i giovani, verso le nuove generazioni, così come era severo con tutta la classe dirigente e politica attuale. Diceva spesso che la politica oggi è debole: è una politica senza una visione non è in grado di risolvere i problemi. Vorrei ricordarlo come un politico capace di farsi ascoltare, anche nei momenti più difficili, un uomo che ha lasciato fortunatamente un patrimonio di valori, di storia, di scritti e di libri; un riferimento per tutti. Abbiamo bisogno, oggi più che mai, più di ieri, di ritrovare e di scommettere sulla politica, quella con la P maiuscola. Abbiamo bisogno di un pensiero politico alto, di una visione per oggi e per domani; abbiamo bisogno di luoghi di discussione e di confronto. Solo così svolgeremo bene il nostro ruolo, anche oggi, da parlamentari, e la nostra funzione nella società. Signor Presidente, c'è bisogno di una cultura riformista di svolgere oggi, con grande senso di responsabilità, questo ruolo. Lasciamo, a nome del Gruppo Italia Viva, le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla moglie Enza, al figlio Antonio e ai suoi adorati nipoti. Perdiamo un grande uomo, ma fortunatamente ci rimane un grande patrimonio culturale. Speriamo davvero, con gli stimoli che possiamo dare da questo importante luogo di discussione e di confronto politico, di invitare le nuove generazioni a leggere i suoi libri, a riflettere e ad approfondire, come è giusto che sia. *(Applausi)*.

anche il Gruppo Fratelli d'Italia rende omaggio a Emanuele Macaluso, che è scomparso a quasi poche ore prima che ricorresse il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano (che credo sia proprio nella giornata di domani, in ricordo di quando alcuni, con Nicolino Bombacci e Antonio Gramsci, fondarono a Livorno il Partito Comunista Italiano da una scissione del Partito Socialista). Macaluso era e nasceva come comunista in anni difficilissimi, con uno spirito ribelle e combattente, ovviamente attento, come allora lo erano i comunisti, ai bisogni sociali e alle lotte operaie e sindacali. Nel contempo, aveva una straordinaria vitalità intellettuale, che mantenne fino all'ultimo giorno della sua esistenza, consapevole come pochi che l'uomo è soprattutto una fucina di idee e vive in quanto esprime le proprie. Lui queste idee voleva comunicarle a tutti e da giornalista le scriveva e le ha scritte sino alla fine. Ricordiamo così Macaluso, che poi divenne con Napolitano uno degli spiriti e dei *leader* dei miglioristi all'interno del Partito Comunista Italiano. E come gli altri miglioristi riuscì poi ad evolvere e a rompere la solidarietà con l'Unione Sovietica. Forse potremmo dire che avrebbe dovuto farlo prima: sicuramente; altrettanto certamente possiamo dire, però, che l'ha fatto prima di tanti altri. Della sua figura ricordiamo l'aspetto più significativo, che ci fa capire chi era, quando da segretario regionale del Partito Comunista, anche su indicazione di Togliatti, decise di varare un Governo il Governo Milazzo, in cui il Partito Comunista votò assessori espressione del Movimento Sociale Italiano.

Ebbene, quella fu l'unica occasione in cui esponenti del Partito Comunista Italiano - parlo del 1958 - votarono esponenti di Governo della Destra di allora, del Movimento Sociale Italiano. Non c'è altro episodio nella storia italiana. Ma quell'episodio, realizzato da Macaluso in sintonia con Nino Buttafuoco (che fu anche il mio maestro politico), dimostra il valore di quella e di altre personalità che fanno parte della nostra storia comune.

...*dimostrando in tal senso il suo valore e la sua personalità. In conclusione, nel ricordarlo come parte della nostra comune storia italiana comune storia italiana e di questo Parlamento, rammento quanto scrisse in un libro per spiegare ai nuovi, ai riformisti, che non potevano rompere del tutto le proprie radici nel comunismo. Questo vale per tutti.

Questo vale ovviamente per i partiti e per i protagonisti di allora, ma vale anche per la nostra storia, non solo per la storia della Repubblica italiana, che è una storia recente, ma per la storia millenaria della nazione italiana.

Signor Presidente, la ringrazio per le sue parole. È per me sinceramente un'emozione ricordare Macaluso, che ho conosciuto ormai molti anni fa. Sono consapevole della mia inadeguatezza. Ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto, anche per il ricordo di un'esperienza politica assolutamente unica, come quella di Milazzo ricordata ora. È impossibile riassumere la sua esperienza: una grande personalità, che ha segnato la storia del nostro Paese, della politica e della cultura italiana. Figlio di una famiglia operaia, sindacalista della CGIL, poi dirigente di primissimo piano del PCI, direttore de «l'Unità», pubblicista, uomo di cultura. Sono Di Vittorio prima e Togliatti poi coloro che valorizzano e investono sulla qualità di Macaluso e sulla sua grande intelligenza; è un protagonista assoluto, è un grande comunista italiano. Ha fatto bene lei, signor Presidente, a sottolinearlo. In una pubblicazione di

il suo PCI nasceva da una condizione sociale forse incomprensibile alle nuove generazioni e che gli è rimasto dentro al cuore, perché ha segnato la sua vita e financo la sua vecchiaia. Un uomo convinto di essere stato un protagonista e un costruttore di un grande percorso politico: il partito nuovo di Togliatti. Stringe un rapporto molto stretto con Berlinguer, poi con Napolitano, tra gli altri, e ha sempre in testa l'idea nazionale, l'idea della Nazione, la via italiana. Su questo si potrà riflettere proprio in questi mesi. Chiunque lo ha conosciuto ne ha apprezzato, oltre all'intelligenza, certamente anche la straordinaria passione politica, che - come è stato detto - non è mai venuta meno, nemmeno negli ultimi giorni. come un insieme di valori, come un progetto politico e una visione del mondo; essa è stata per lui il modo di essere moderno, libero e, nello stesso tempo, profondamente legato alla sua comunità, come ha avuto modo di sottolineare Castellina oggi in un articolo, che ricorda che egli fu uno dei pochissimi dirigenti che, all'indomani dell'espulsione delle persone de «il manifesto», continuasse a incontrarli, a salutarli, ad apprezzarli. Si è costruito non sulla base di un impianto ideologico; ma, dalla lotta a favore dei contadini alla lotta alla mafia, si è costruito nel processo sociale reale. Un riformista,

e senza nessuna reticenza. Era un uomo libero perché forte e saldo nei contenuti e dallo spirito critico, senza mai abbandonare la sua comunità. Credo che ci mancherà

Macaluso non ha mai rinunciato a porre un problema: bisogna ricostruire la sinistra di massa.

avere spirito critico, misurarsi con le grandi novità che saranno il fondamento di una sinistra moderna come è stato detto a proposito della metafora del pozzo - senza mai dimenticare le radici profonde che sono rappresentate magnificamente anche nelle contraddizioni e nella vita straordinaria di Emanuele Macaluso.

ieri mattina presto, prima che fossimo in Aula, abbiamo ricevuto la telefonata del senatore Ugo Sposetti che comunicava al Gruppo Partito Democratico la scomparsa di Emanuele Macaluso. Il nome e la figura di Emanuele Macaluso sono molto più del lascito della sua attività parlamentare, che svolse a partire dagli anni Sessanta, prima alla Camera e poi qui al Senato. anni di tumultuose trasformazioni egli fu sempre analista lucido e mai dogmatico. Furono anni di rivendicazioni e di conquiste sociali di cui egli fu protagonista da dirigente politico di primissimo piano del Partito Comunista Italiano, una forza sociale e un gruppo dirigente senza il cui apporto decisivo e sostanziale noi non avremmo la Costituzione della nostra Repubblica così avanzata come la conosciamo oggi. Emanuele Macaluso spesso rimarcava La sua scomparsa a quasi cento anni avviene nei giorni del centenario della nascita del Partito Comunista Italiano e della scissione drammatica di Livorno. In tutta la sua vita politica Macaluso si è battuto per l'unità della sinistra e per le ragioni storiche dell'incontro tra le forze democratiche e riformiste. Lo ha fatto nei passaggi più duri della nostra vicenda repubblicana, come quello segnato dal terrorismo, o successivamente negli anni dello scollamento sempre più forte tra società e istituzioni, che ancora adesso attanaglia in una crisi la nostra democrazia. Per tanti di noi, che sono stati giovani militanti negli anni Ottanta, quella di Macaluso era una delle figure del leggendario, ai nostri occhi, gruppo dirigente comunista. da Togliatti nel 1956, anno paradigmatico, per contribuire a costruire un partito popolare radicato nell'urgenza dei nuovi bisogni sociali. Veniva dalle lotte concretissime del sindacato ed era stato voluto da Di Vittorio alla guida della camera del lavoro di Caltanissetta e poi del sindacato nell'intera isola. Era nato da una famiglia povera povera nella terra poverissima delle solfatare in Sicilia. Nella sua vita di militante politico ed intellettuale ha sempre incarnato gli ideali di emancipazione e di giustizia sociale che lo hanno portato da ragazzo a scegliere di stare dalla parte di braccianti, operai e diseredati. Quando penso a Macaluso penso ai morti di Portella penso ai morti di Portella della Ginestra, ai mitra della mafia contro le lotte dei braccianti e dei minatori, alla lotta per la riforma agraria, per dare la terra a chi la lavorava. Macaluso è stato tutto questo e innumerevoli altre cose, perché ha vissuto tante vite in un tempo intensissimo e duro. Giornalista e polemista di rara intelligenza e statura politica, fu al fianco di Berlinguer da dirigente politico. A lui toccò in sorte di essere direttore de «l'Unità» nei giorni terribili della morte di Berlinguer, sapendo lasciare dalle pagine del giornale la testimonianza storica di un moto emotivo enorme, di un lutto collettivo nazionale. I suoi interventi sulla questione sociale e sulla questione meridionale parlano ancora oggi con forza a chi voglia ricostruire una cultura politica di Fu comunista e riformista, rivendicando il nesso tra le due cose nella vicenda storica italiana. Fu strenuo garantista, in dialogo serrato e fecondo con Leonardo Sciascia; fu europeista, socialista, sempre; fu uomo di assoluta passione politica e rigore morale. Di Emanuele Macaluso ci sono tante e bellissime immagini e, tra queste, quelle che lo ritraggono con il presidente Giorgio Napolitano. Il loro sodalizio umano e politico è durato tutta la vita. Emanuele Macaluso è stata lucida coscienza critica della sinistra e della Repubblica italiana. Non ha mai smesso di denunciare il pericolo della mancanza di partiti strutturati e radicati, di una politica debole, catturata da poteri forti. Non ha mai smesso di denunciare il pericolo della mancanza dell'autonomia della politica, il pericolo del populismo e dell'antipolitica come tradimento delle giuste istanze dei più deboli. signor Presidente - un grande italiano, uno degli interpreti più lucidi e migliori della grande lezione del nostro Novecento e continuerà ad essere riferimento fondamentale per chi crede nella democrazia e nel nostro Paese. Signor Presidente, sono grato infine perché so che il Senato della Repubblica italiana domani, parteciperà ai funerali di Emanuele Macaluso che avranno luogo a Roma. *(Applausi)*.

un gigante dell'analisi politica oltre che un gran galantuomo, non è morto ieri: è morto nel 1989 con la caduta del muro di Berlino, non perché sotto le macerie del muro di Berlino rimase schiacciato quel che restava del suo mondo

la politica della visione e delle radici che programmano un futuro. Questa era la vera identità di Macaluso. Era un uomo politico formatosi nei tempi in cui la politica aveva un valore e una dignità, in cui assumeva un primato. per uno come me, anticomunista totale, non è stato per niente difficile avere un rapporto profondo con una personalità del genere, come non lo è stato con altri testimoni di altre culture politiche, ma di quell'epoca, come Francesco Cossiga e Rino Formica, tanto per citare le tre culture politiche che hanno animato, nel bene e nel male, la storia della prima Repubblica: tutte personalità che credevano nel primato della politica, espresse da un mondo che non esiste più, ma che non hanno rinunciato a testimoniare l'esistenza in vita di quel mondo, a rendergli onore. A dire dire la verità Macaluso non era il perfetto *testimonial* del Partito Comunista: era in minoranza nel PC, era amendoliano, era migliorista. Era, come avete ricordato in molti ed è stato giusto ricordarlo, un garantista, in linea e in perfetta sintonia con un altro galantuomo siciliano come Leonardo Sciascia e, di conseguenza, di conseguenza, aveva rapporti profondi con i radicali, cosa inammissibile allora per un comunista togliattiano integrale. Era così perché era un uomo libero e la sua libertà di uomo gli costò un processo non soltanto in sede giudiziaria, ma anche in sede politica. Mancò poco che fosse cacciato dal Partito Comunista Italiano per aver commesso la colpa grave di essersi innamorato di una donna sposata. Erano altri tempi, il moralismo allora allignava più nei ranghi del Partito Comunista che in quella della Democrazia Cristiana, paradossalmente, la morale era doppia, ma questo è un altro discorso. Credo che la figura di Macaluso vada ricordata per la sua coerenza e per la sua libertà estrema. Macaluso non ha mai rinnegato la sua storia di uomo, la sua storia politica, non ha mai rinnegato il comunismo in un'epoca in cui tutti rinnegano tutto, ha sempre cercato di spiegare in un'epoca in cui nessuno riesce a spiegare più nulla. È morto tenendo alta la dignità e l'importanza della l'importanza della politica. È morto sull'attenti come la sentinella trovata pietrificata a Pompei dopo l'eruzione del Vesuvio; sull'attenti perché nessuno - nel caso di Macaluso, non un uomo, ma la storia - aveva sciolto la consegna che aveva ricevuto. *(Applausi)*.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è per me un onore ricordare in questa Aula, a nome del partito a cui appartengo, Emanuele Macaluso, morto ieri all'età di novantasette anni. Mi piace ricordarlo innanzitutto per quanto ci ha appena lasciato. Solo poche settimane fa aveva terminato la revisione delle bozze del suo ultimo libro «Comunisti a modo nostro», che uscirà a breve. È frequente che le menti più lucide e più brillanti, proprio perché tali, rimangano efficienti fino all'ultimo ed Emanuele Macaluso, licenziando il suo ultimo libro alla straordinaria età di ci consente di continuare il dialogo con lui, pur dopo la sua scomparsa. La quarta di copertina ci racconta che a cento anni dalla fondazione del Partito Comunista, Emanuele Macaluso e Claudio Petruccioli ne ripercorrono sviste e svolte epocali, ricordando le conquiste sociali di cui fu promotore e ipotizzando strade alternative che l'Italia avrebbe potuto imboccare per scongiurare il declino politico e culturale del Paese. Macaluso si iscrive con coraggio al Partito Comunista quando in Italia è ancora al potere il fascismo e per tutta la sua vita rimarrà fedele alla sua scelta iniziale. Ho detto fedele e non coerente perché l'arte della politica impone di adeguare il proprio pensiero e le proprie azioni ad una variabile non controllabile qual è il divenire delle società umane. Macaluso fu tra coloro che intuirono la necessità di rendere la sinistra italiana parte la dottrina del marxismo come dottrina dello Stato aveva terminato ed esaurito la sua spinta propulsiva.

non già di abbattere il capitalismo, ma di contrastarlo per attenuarne la tendenza a travolgere la persona umana e farne solo un fattore del mercato. Avevamo ed abbiamo bisogno di persone come lui, qualunque sia lo schieramento politico in cui ci riconosciamo perché la democrazia è nella sua ultima essenza confronto per giungere ad una sintesi che sia la migliore per il Paese. Emanuele Macaluso, con la sua figura, ci ricorda che in politica esistono avversari e non già nemici ed è di questa idea che oggi l'Italia ha bisogno più che mai. mai. Addio senatore Macaluso, che noi tutti si possa rappresentare degnamente la tua eredità morale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con emozione che oggi ricordiamo il senatore Macaluso, storico dirigente del Partito Comunista Italiano, sindacalista, giornalista e direttore de «l'Unità». Ricordare e commemorare in quest'Aula una figura come quella di Macaluso non è affatto semplice. Possiamo dire che il suo percorso umano, civile e politico reca impressi i caratteri di quella straordinaria crescita democratica che ha consentito al nostro popolo di liberarsi dal fascismo, di dotarsi di una Costituzione rispettosa degli originari e inviolabili diritti della persona, di progredire nel benessere economico e nella solidarietà sociale. Andreotti a parte, la vita di Emanuele Macaluso è rinchiusa per me in una frase che lui disse sulle colonne de «L'Espresso». Disse di esser diventato comunista per ribellione. In questa frase c'è tutto il senso delle scelte di una vita e io desidero in questa sede ricordare il suo impegno politico di figlio del Sud, maturato da giovanissimo, motivato dalla volontà di emancipazione dei più deboli e di tutela dei lavoratori, sviluppandosi nella CGIL e nel Partito Comunista Italiano con iniziative su eventi coraggiosi e difficili, chiamato da Giuseppe Di Vittorio a soli ventitré anni a dirigere in Sicilia il sindacato dei braccianti qualifica oggi abusata da politici di seconda fila per lucrare posizioni di potere spesso non meritate *(Applausi) -*, in anni in cui ai comizi di Girolamo Li Causi la mafia rispondeva con le bombe e con i mitra. Macaluso è stato un protagonista della storia repubblicana e ha contribuito, da dirigente politico e da intellettuale, alla crescita democratica del Paese. Un grande siciliano, ma anche un grande meridionalista, che si sforzava di mettere nella giusta luce la sua Sicilia e l'intero Mezzogiorno; un Mezzogiorno che a suo parere avrebbe dovuto usare persino la crisi come occasione per ripensarsi e scommettere sull'innovazione, sul cambiamento necessario, sul bisogno di scrollarsi di dosso vecchie mentalità e indolenze culturali; un Sud, secondo Macaluso, che doveva sentire anche il dolore sociale, la fatica di vivere, la domanda persino disperata di lavoro di quelle giovani generazioni ingabbiate nei circuiti lividi della precarietà. Ammoniva tutta la politica a tornare ad investire quantitativamente e qualitativamente su formazione, educazione, cultura e ricerca recuperando capacità di ascolto delle delle competenze e delle passioni di chi vive nella scuola e nell'università. Signor Presidente, colleghi, come ha scritto oggi un suo vecchio compagno ricordando Macaluso, la storia del Partito Comunista Italiano è una storia nobile, ma a tratti contraddittoria, che però ha segnato per intero la nostra cultura democratica anche in momenti in cui il coraggio di una certa dirigenza di quel partito, della quale Macaluso era parte integrante, mancò l'occasione di smarcarsi per tempo dal cappio ideologico del regime sovietico e che probabilmente avrebbe cambiato il corso della nostra storia recente, magari non ostacolando quell'alternativa di sinistra che negli anni Settanta l'Italia avrebbe potuto sperimentare per uscire da un regime democratico cristiano ormai decotto, come la vicenda di tangentopoli e il tramonto della Prima Repubblica hanno dimostrato Tuttavia altri diranno e scriveranno più compiutamente sulla figura di Emanuele Macaluso e su quegli anni contraddittori, magari sfruttando l'onda del centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano. Oggi sentiamo Oggi sentiamo di essere grati a quest'uomo, a questo dirigente politico, sindacalista e giornalista che, con intelligenza, passione, curiosità e coraggio, ha attraversato con lealtà la storia italiana, dando un grande contributo alla crescita civile del nostro Paese. Alla famiglia vanno le mie condoglianze e quelle di tutti i senatori del MoVimento 5 Stelle.

Grazie

Signor Presidente, il Governo ha trasmesso al Parlamento la relazione che illustra l'aggiornamento del Piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine rispetto a quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020, già modificato, per il solo 2020, con la relazione approvata dalle Camere il 26 novembre scorso. La relazione in esame è adottata ai sensi dell'articolo 6

dall'obiettivo di medio termine siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il Piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine. È opportuno ricordare che nell'anno 2020 sono state approvate dalle Camere autorizzazioni allo scostamento dal Piano di rientro per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19. In premessa, il Governo richiama sia la decisione della Commissione europea di applicare la cosiddetta *general escape clause* del patto di stabilità e crescita sia la raccomandazione, rivolta dalla medesima Commissione agli Stati membri, di mantenere, anche per il 2021, una intonazione espansiva della politica di bilancio. Il Governo evidenzia preliminarmente che, a causa delle ulteriori restrizioni introdotte a dicembre per il contenimento dell'epidemia e del tempo necessario per completare la campagna di vaccinazione, i settori a maggiore intensità di contatti sociali continueranno a essere influenzati negativamente dalla pandemia. Pertanto, le stringenti misure sanitarie richiedono di essere accompagnate da interventi di sostegno e ristoro di entità nettamente maggiore rispetto a quanto preventivato nella legge di bilancio 2021. In particolare, il Governo ha intenzione di adottare misure riguardanti nuovi stanziamenti a tutela del lavoro: aumento del sostegno alle autonomie locali, incremento delle risorse per la Protezione civile e le forze dell'ordine, ulteriori risorse per il settore sanitario (in particolare nel quadro della campagna di vaccinazione e del trattamento di pazienti affetti da Covid-19), risorse aggiuntive destinate al sistema dei trasporti pubblici, rimodulazione temporale dell'invio delle cartelle esattoriali e una serie di misure a favore Il Governo richiede, quindi, per il corrente anno, l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche; 35 miliardi di euro in termini di fabbisogno; di 40 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza; di 50 miliardi di euro, in termini sempre di saldo netto da finanziare, in termini di cassa. Richiede, inoltre, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento per i maggiori oneri derivanti dal servizio del debito fino a 200 milioni annui nel biennio 2022-2023; 300 milioni di euro annui nel biennio 2024-2025; di 400 milioni di euro annui nel 2026-2027; di 500 milioni di euro annui nel 2028-2029; di 600 milioni di euro nel 2030 e di 700 milioni di euro a decorrere dal 2031. Tale scostamento ridetermina, quindi, sia il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1 della legge di bilancio 2021, sia l'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. A differenza di quanto riportato nella precedente relazione al Parlamento, quella in esame non indica espressamente i nuovi valori comprensivi del ricorso al maggiore indebitamento richiesto, dell'indebitamento netto della PA per il 2021, né in termini assoluti né in percentuale di PIL, e del debito pubblico rispetto al PIL. Considerando i valori indicati nella NADEF 2020, nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2021-2023 e, da ultimo, della nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio 2021-2023, per effetto dell'autorizzazione richiesta, l'indebitamento netto della PA aumenterebbe in valore assoluto a circa 105,6 miliardi di euro, con una incidenza rispetto al PIL pari a circa l'8,8 per cento. Al riguardo, ricordo all'Aula che il Ministro, in audizione, ha confermato questi dati. La relazione evidenzia inoltre che, considerata la natura temporanea degli interventi, resta sostanzialmente confermato che dal 2022 il percorso di rientro verso l'obiettivo di medio termine, già indicato nella NADEF 2020, è risultante dalla applicazione della legge di bilancio 2021-2023. Da ciò sembrerebbe discendere il carattere sostanzialmente neutrale dello spostamento richiesto in termini di saldo di bilancio strutturale. Per quanto attiene al debito, in valore assoluto, l'incremento dovrebbe risultare dell'ordine di 35 miliardi di euro per l'anno 2021, corrispondente all'aumento richiesto dal fabbisogno. Per eventuali approfondimenti, si rimanda alle note del Servizio studi e bilancio della Camera e del Senato. *(Applausi)*.

la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento di bilancio e autorizza il piano di rientro all'indebitamento è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Le proposte di risoluzione riferite alla relazione dovranno essere presentate

ha affrontato - in termini forse non tanto politichesi, molto duri e diretti - un tema sul quale credo quest'Assemblea debba assolutamente riflettere, posto che tutti sappiamo che oggi siamo favorevoli allo scostamento di bilancio. Sostanzialmente il senatore Monti dice che diviene importante porsi con urgenza il problema di quanto abbia senso continuare a ristorare con debito le perdite di molte attività per le quali sarebbe meglio che lo Stato favorisse la ristrutturazione o la chiusura.

a dove finiranno questi ristori, che non sono assolutamente sufficienti - e tutta l'Assemblea è d'accordo, destra e sinistra, sull'affrontare questo ulteriore scostamento di bilancio e quindi mi riferisco soprattutto al mondo del commercio e dei pubblici esercizi, credo che si debba necessariamente riflettere (lo dico da liberista, cioè, da persona che crede nel libero mercato) sul fatto che forse questa concorrenza senza regole - mi riferisco in modo particolare a quella famosa liberalizzazione delle licenze voluta da Bersani qualche problema lo sta dando. Mi spiego meglio. Ci sono una serie di attività che proprio non ce la fanno più. La concorrenza che ha portato verso il basso la qualità dei servizi e dei beni,

seconda riflessione. Sappiamo che una parte dei ristori va a sostenere la cassa integrazione. Ebbene, vorrei dirvi cosa è successo a ottobre, un dato che è stato diffuso dal dipartimento del *welfare* di Zurigo. Si tratta di una notizia molto interessante: a ottobre 2020, ben 26 assistenti di volo della compagnia Swiss International Air Lines lavoravano per il tracciamento dei contatti del Covid. Cosa voglio dire con questo? Che l'Italia è estremamente indietro, che bisogna fare un'operazione culturale fortissima perché ci saranno tutta una serie di mestieri che scompariranno e noi continuiamo, invece, a finanziare la cassa integrazione prestare attenzione a che cosa? L'ho chiesto più volte: a quella riqualificazione del capitale umano che in certi casi è assolutamente possibile. La testimonianza di questi 26, due dei quali

fu ridicolizzato, gli fu detto che non era il caso, che era troppo, che era una cifra astronomica. Ancora nella discussione di ieri, un collega della maggioranza ha detto che il senatore Salvini giocava al Fatti i debiti conti, oggi ci troviamo a cavallo tra il 2020 e il 2021, in condizione di aver fatto scostamenti

la Lega e il suo *leader* Salvini dissero che c'era bisogno di cominciare a mettere subito sul tavolo 100 miliardi di euro, per poi verificare esattamente le situazioni. Così non è stato e ci troviamo adesso, a distanza di quasi un anno, quasi alla terza ondata pandemica, con i *lockdown* che si alternano a situazioni di apertura, ad approntare un altro scostamento di ben

quando sarà ora di prendere delle decisioni e se faremo come è successo ieri, avanti e indietro con le compravendite, mentre fuori la malattia prosegue, le attività chiudono, ci sono i fallimenti,

non va bene. È stato detto che non c'è la preveggenza (se fossimo preveggenti non saremmo qui), ma c'è il buon senso e c'è l'intelligenza, che non deve mai sostituirsi alla intellighenzia, che è altra cosa.

Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la grave crisi scaturita dalla virulenza della pandemia globale in corso sta facendo traballare gli assetti produttivi e, quindi, anche la rete di protezione sociale,

un'ulteriore crisi che ha un nome e un cognome e che, per insulsi giochi di potere, ha colpito in modo sconsiderato un popolo in ginocchio; un popolo che lotta per affrontare i mille problemi che vive quotidianamente

un grandissimo risultato che non può prescindere da forze politiche compatte, con il capo chino a lavorare incessantemente. Il popolo italiano non può aspettare, non può sopportare che si stia a giocare con i reali problemi che si stanno vivendo ora, in questo momento. Il debito concesso deve essere utilizzato in maniera efficiente e rapida, come l'Italia dimostrò di saper fare con i fondi del piano Marshall per la ricostruzione del secondo Dopoguerra. scossone anche per l'agricoltura, che è al secondo cambio di Ministro, in una legislatura caratterizzata da improvvise, quanto immotivate picconate; tentativi di scalare un monte ora da destra ora da sinistra, ma decisamente troppo alto da scalare. Ma il nostro presidente Conte, con la nostra lealtà e il nostro sostegno, riuscirà a portare a compimento un lavoro iniziato e condotto con grande perizia. Dati i fatti, purtroppo, al Ministero dell'agricoltura ora languono importanti provvedimenti provvedimenti per il ristoro di molte attività, come il *bonus* ristorazione, voluto dall'ex Ministro, che non è ancora arrivato agli operatori: parliamo di 600 milioni di euro del decreto agosto a sostegno della filiera agroalimentare per gli acquisti fatti da ristoranti, pizzerie, *catering*, mense, agriturismi e alberghi. Queste imprese hanno bisogno di una politica che abbia come unico obiettivo l'uscita dalla crisi e la garanzia di adeguati sostegni con tempistiche celeri e una burocrazia più snella ed efficace. È indispensabile un lavoro costante; insomma, Ministri e parlamentari al lavoro e non impegnati in inutili balletti. Intanto la vera crisi, quella della pandemia, sta dimostrando di non voler allentare la morsa. I tempi per venirne fuori non sono brevi e quindi si è resa necessaria un'ulteriore rivisitazione dei conti. Abbiamo l'urgenza di dare risposte a quelle attività maggiormente colpite dalle restrizioni, in particolare i settori della ristorazione, dello spettacolo, del turismo e dello sport, nuovi stanziamenti anche per la tutela del lavoro alle amministrazioni territoriali, alle Forze dell'ordine, al sistema di Protezione civile, al sistema dei trasporti pubblici, alla sanità, alla rimodulazione dei tempi di invio delle cartelle esattoriali; misure che si traducono in un fabbisogno di risorse maggiore di quanto preventivato nella legge di bilancio. Eccoci, quindi, ad approvare lo scostamento necessario. Oggi al voto vi è l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento per 32 miliardi di euro netti; momento delicatissimo, in cui anche il lavoro sul *recovery plan* italiano è in corso. La politica ha il dovere di portare avanti questo grande impegno, che l'Italia intera, coesa, deve mettere in atto.

Tre sono le ricette per affrontare il debito:

fare debito, poi si vedrà; intanto facciamo il Presidente della Repubblica. La seconda è la ricetta Monti, ribadita ieri: cupa tristezza fiscale. La ricetta del centrodestra: l'economia è sensazione, è voglia di migliorare.

Voi che fate? Il *cashback* per tre miliardi. Alleviamo tutti fighetti che pagano tre euro con la carta, ma non distinguono una mucca da un toro. *(Applausi)*. Stornate questi soldi e metteteli ai ristori. Quei fighetti, poi, prendono il reddito di cittadinanza e aspettano la pensione. Il sistema Italia è così piazzato. Noi abbiamo 3.500 miliardi di debito (2.600 pubblico certificato); due finanziarie in fase di digestione (da 40 miliardi debiti commerciali per 50 miliardi di euro; scostamenti - con oggi - per 160; crediti fiscali dei contribuenti quantificati in 50

di euro e deve essere usato solo in conto capitale, non in sostituzione, da restituire direttamente o indirettamente, da realizzare a *step*. L'Italia in questa situazione - e voi lo sapete - non è neanche in grado di progettare le opere. Ci sono poi altri debiti, secondo me nascosti, ma sto indagando e la prossima volta riferirò. Ci sono i prestiti bancari, mutui e fidi, per 2.300 miliardi, che sono aumentati a seguito delle garanzie dello Stato e anche per le giuste proroghe del rimborso delle rate. Abbiamo in attivo 1.900 miliardi di depositi; qualcuno pensa di espropriarli, ma sostengono i prestiti. Le azioni e obbligazioni ammontano a 2.300-2.500 miliardi (sono cifre variabili). Gli immobili oggi sono in crisi nera - la verità è questa - escluse certe situazioni.

chi è sovrano della moneta non fallisce: ne può stampare quanta ne vuole. L'Italia non può, perché è nell'euro. Non dico di uscire, perché non è possibile, ma la ricetta, non potendo stampare, è una sola, quella che ho indicato in partenza: produrre ricchezza. Non c'è altra scelta. Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, senatori e senatrici, stiamo vivendo giorni molto particolari per il nostro Paese: incertezza, paura e rabbia sono i sentimenti che prevalgono nei cittadini dopo un anno di dolore e di sacrifici causati da questa terribile pandemia. A questi si aggiunge chi ha spregiudicatamente deciso di far nascere una crisi di Governo in un momento così delicato. Oggi non è tempo di demolire ma di costruire. È il momento di dimostrare dignità, responsabilità, rispetto dei principi morali e personali. Obbligo morale è avere come unico, imprescindibile obiettivo quello di lavorare a testa bassa per le priorità del popolo italiano, mettendosi al loro servizio. Serve impegnarsi notte e giorno per continuare a trovare soluzioni ai problemi del Paese. All'Italia non serve chi non vuole risolverli e preferisce in questo momento crearne altri; non serve a questo Paese chi, in questo tragico frangente, ha scelto gli interessi propri e di partito e di giocare con il futuro della vita degli italiani. Come già indicato da tutti gli esperti, la curva dei contagi non è rassicurante. Saremo ancora costretti sulla strada delle misure restrittive, dolorose ma inevitabili. Grazie all'arrivo dei vaccini, speriamo di poter allentare presto le eccezionali misure di contenimento della pandemia. La diffusione dell'epidemia preoccupa preoccupa per la tenuta del Sistema sanitario nazionale e ha richiesto l'adozione di provvedimenti difficili da parte del presidente del Consiglio Conte e del suo Esecutivo, che noi sosteniamo convintamente. Gli italiani sono chiamati a lottare, a resistere, ad affrontare importanti sacrifici. Nei loro confronti, per onorare il ruolo che ricopriamo con le mani libere attraverso le nostre scelte, dobbiamo dimostrare grande senso di responsabilità, umiltà e rispetto; scelte che inevitabilmente hanno ripercussioni su attività produttive e operatori economici, su lavoratrici e lavoratori, su intere famiglie, verso cui abbiamo l'obbligo morale di dare sostegno immediato. *(Applausi)*. Dobbiamo dare risposte a chi chiede supporto.

una cifra ingente di risorse messe in campo in un solo anno per evitare una grave depressione economica e favorire la ripresa celere. sono crisi di Governo, personalismi e scelte irresponsabili che debbano rallentare le azioni a sostegno della Nazione. Le priorità fin dall'inizio della pandemia sono la tutela dei cittadini e il sostegno alle attività produttive e ai lavoratori. ai lavoratori. In uno scenario economico e sociale che non ha precedenti nella nostra storia, nel momento più difficile della storia della Repubblica, bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, senza alcun indugio. Continuiamo con gratitudine e orgogliosi a sostenere il presidente Conte e la linea di Governo assunta. Lo facciamo anche votando a favore dello scostamento di bilancio e del conseguente decreto-legge ristori. Vanno cercati Vanno cercati non onori e ringraziamenti nel fare la cosa giusta, ma solo la dignità, che si può indossare e che è l'unico vero premio a cui si deve tendere nel fare il proprio dovere. Signor Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, sono state giornate convulse quelle che abbiamo vissuto in questa settimana, in un momento così delicato e particolare per il Paese. Da un anno il futuro del nostro Paese, per la crisi sanitaria ed economica, è incerto. Ieri abbiamo assistito in quest'Aula all'ennesimo voto di fiducia; possiamo dire forse all'ennesimo voto al fotofinish - è finita infatti in questo senso - ottenendo il Governo una semplice maggioranza aritmetica. È chiaro che tutto è legittimo costituzionalmente e che in questo momento l'aritmetica è dalla parte del Governo, ma non lo è sicuramente la politica. Quella attuale è una maggioranza solo apparente che si mantiene in vita per accanimento terapeutico, direi. Per ironia della sorte, proprio in quest'Aula a poche ore dal voto di ieri, si affronta un provvedimento molto importante, quello dello scostamento di bilancio, per il quale la maggioranza e il Governo non hanno i numeri sufficienti a favore.

debito sulle future generazioni. Si tratta di interventi, quelli sullo scostamento di bilancio e quelli che verranno anche per il decreto-legge ristori, sicuramente meritevoli in un momento particolare per il Paese. Questo Governo oggi fa fatica a raccogliere il consenso, anche all'interno della sua stessa maggioranza. Perciò il paradosso oggi si manifesta e diventa lampante. Se non ci fossero parlamentari e le forze di centrodestra, come il Gruppo parlamentare di Forza Italia, che sta sostenendo questi provvedimenti in favore del Paese, in favore dei lavoratori autonomi, delle partite IVA e dei commercianti, oggi il Governo non avrebbe i numeri

a essere penalizzata. Tirando le somme, è vero che non si può assolutamente negare in questo momento un voto favorevole allo scostamento di bilancio, ma è pur vero che non possiamo condividere il *modus operandi* di chi ancora si ostina a suonare il violino su una nave che affonda.

Signor Presidente, nel poco tempo messo a disposizione su questo tema, che meriterebbe una riflessione profonda, mi soffermerò solo su alcune parti, relativamente all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine e al conseguente scostamento di bilancio. Nella relazione al Parlamento comunicata il 15 gennaio 2021 leggo, all'ultimo paragrafo («Finalità del provvedimento e piano di rientro»), sono previsti nuovi stanziamenti per interventi a favore della dotazione di ulteriori risorse per le Forze dell'ordine e per il sistema di Protezione civile. Questa relazione è molto vaga ed è stata scritta secondo macroargomenti. Vorrei porre l'attenzione su questo argomento, perché la Lega è ovviamente vicina alle Forze dell'ordine, che hanno bisogno di un maggior sostegno, anche economico, ed è favorevole all'impegno di risorse a favore della Protezione civile.

qual è l'intento di questo Governo: continuare a portare avanti l'invasione di clandestini. La priorità va agli italiani. Sapete bene, caro Governo, quanto siano in difficoltà e quanto abbiano bisogno di aiuto. Spesso ci rispondete che manca il tempo. Come calendarizzare quindi con rapidità eventuali ristori ed eventuali provvedimenti che vadano a favore degli italiani?

Il tempo è stato sacrificato per smontare i decreti Salvini. Quindi, mi raccomando e mi auguro

perché si è visto esautorato e ha visto sacrificata la democrazia, che da quando voi siete al Governo non viene più portata avanti.

Grazie Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, si rende necessario un altro scostamento di bilancio per una cifra considerevole perché c'è bisogno di nuovi ristori. È doveroso assicurare agli operatori economici, ai settori produttivi e alle categorie di cittadini in affanno una ulteriore iniezione di liquidità e sono convinta che Governo e Parlamento continueranno a sostenere lo sforzo del Paese, piegato dalla pandemia, ma soprattutto incerto davanti a un futuro che è diventato difficile da immaginare. Il futuro non è fatto, però, esclusivamente di cose. Perciò, anche se la parola «cultura» non compare neppure nella relazione al Consiglio dei ministri su quest'ultimo scostamento, è di cultura che voglio parlare nei pochi minuti a disposizione e dei ristori di cui ha bisogno questo settore che, oltre all'irriducibile valenza spirituale, ne possiede anche una materiale e - al contrario di quanto dicono le letture distorte e opportunistiche correnti - sta letteralmente agonizzando. (PNRR) 8 miliardi sono destinati alla cultura: 2,7 andranno al patrimonio culturale per la Next Generation EU; 2,4 al trinomio siti minori, aree rurali e periferie; 2,9 a turismo e cultura 4.0. Non bastano - lasciatemelo dire - e non sono diretti dove è più necessario e urgente. La digitalizzazione, infatti, non è una panacea e la rigenerazione dei borghi e delle periferie non garantisce il funzionamento della rete, delle aree archeologiche, dei musei, degli archivi e delle biblioteche, né salva i centri storici e l'edilizia storica in genere. Non bastano al turismo gli otto miliardi e non bastano alla cultura, che ancora una volta è stata incatenata al turismo, senza capire che ridurla a quello soltanto è una visione miope basata sull'assenza di quei bilanci che, se esistessero, certificherebbero la fallimentare gestione economica del nostro patrimonio culturale. Pensate che persino a Pompei, che pure è il palcoscenico dell'archeologia mondiale, il direttore Osanna certifica che non esiste un tariffario generale che fissi l'importo da corrispondere per le concessioni d'uso per le fotografie, i filmati e le mostre. avviene perché manca a livello nazionale una regolamentazione giuridico-economica al riguardo fuori dalle generiche previsioni del codice Urbani, che però risalgono al 2004. Mentre resta incompresa e insoddisfatta la necessità estrema di investimenti di cui quel settore ha bisogno per non collassare definitivamente, impazza l'idea dei beni culturali come beni esclusivamente strumentali e commerciali da vendere al miglior offerente invece che gestirli con oculatezza. È la mercificazione della cultura - e non la cultura - a essere inscindibile dal turismo. È nell'ottica distorta del mercato che i beni culturali sono sacrificabili e sacrificati oggi dalla stessa amministrazione che la Costituzione chiama per tutelare e valorizzare l'intero ed enorme patrimonio artistico e paesaggistico italiano di cui siamo coeredi, insieme al resto dell'umanità vivente e, soprattutto, alle generazioni future, e, dunque, anche custodi. A divorare quei beni è un turismo incentivato tutt'ora nella prospettiva pre-Covid, sperando cioè che possa tornare a consumare le città d'arte, con milioni di frettolosi avventori affamati di cibo e di emozioni, addestrati a reagire agli stimoli condizionanti del clamoroso - che clamoroso non è del misterioso - che misterioso non è - e dell'irripetibile, che tuttavia si ripete a comando per i fortunati clienti. Il fatto è che si stenta anche in Parlamento e al Governo, qualsiasi esso sia, a riconoscere centralità alla conoscenza e valore strategico alla cultura. Sarà forse anche per questo che, tra i cinque senatori che la settimana scorsa nell'assemblea dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle hanno affidato a un collega della Camera il compito di esprimere una posizione condivisa che chiede un cambio di passo al movimento, quattro sono membri della Commissione cultura? Aggiungo che sono - siamo - tutte e quattro donne. Anche questo è significativo. Sarebbe un delitto ignorare il campanello d'allarme che da quel mondo impazza da ben prima dell'avvio della pandemia. Non a caso esso rimprovera oggi al MoVimento di aver marciato, nel 2016 insieme a chi si opponeva al "sistema Franceschini" di gestione del patrimonio, per poi farsene complice. Sarebbe un delitto anche continuare a disincentivare l'educazione, e cioè a investire nell'ignoranza - e sto parlando di scuola e università - nonché alimentare la retorica deresponsabilizzante della bellezza che salverà il mondo. La bellezza salva il mondo solo se produce nuova bellezza. Allo stesso modo, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura - parlo dell'articolo 9 - per nessun'altra ragione se non perché essa generi nuova cultura. Ben vengano allora gli otto miliardi del PNRR, ma ben vengano, soprattutto, vengano, soprattutto, per stabilire quanto spetti alla cultura e quali iniziative debbano essere finanziate. Ben venga la riaffermazione dei principi in nome dei quali si erogano tali risorse, strumenti per raggiungere uno scopo più alto. Vogliamo chiamarlo bellezza? Sia pure, ma ricordiamoci che non...

Signor Presidente, gentili colleghi, rappresentanti del Governo, ancora una volta quest'Assemblea si appresta ad autorizzare un'importante scostamento di bilancio. Con i 32 miliardi di oggi arriviamo a toccare quota 155 miliardi, una cifra imponente, commisurata tuttavia alla risposta che siamo chiamati a dare al Paese in un momento così difficile. Ancora oggi la discussione tra noi e nel Paese risente indubbiamente della crisi politica che stiamo vivendo, ma su questi temi signor Presidente, cari colleghi - sul futuro del Paese e delle future generazioni non c'è crisi politica che tenga. Di fronte a queste scelte ognuno di noi è chiamato al più alto senso di responsabilità. Certo, dovremo accompagnare questa responsabilità con la capacità reciproca di saperci ascoltare e far diventare questo luogo non soltanto uno spazio nel quale ciascuno pone i propri «si deve», ma dove ognuno ascolta le posizioni degli altri. motivo - e mi rivolgo al Governo - vorrei che sentiste forte la responsabilità della quale quest'Assemblea e il Parlamento tutto vi stanno ancora una volta investendo. Stiamo decidendo di utilizzare risorse che non abbiamo, facendo altro debito; un debito che peserà enormemente sulle nuove generazioni, ma che siamo chiamati a fare per rispondere alle tante istanze che arrivano dai cittadini, dalle continue richieste di aiuto, di sostegno, dall'emergenza e dall'esigenza di dimostrare che lo Stato c'è, soprattutto nei momenti difficili. Stiamo parlando di un debito che non è quello buono cui l'ex presidente della BCE, Mario Draghi, ci ha chiesto di prestare attenzione. È per questo che Italia Viva in questi mesi ha sempre insistito affinché si vada a toccare il nodo centrale della crescita per il nostro Paese, in modo tale che l'ingente debito che oggi stiamo producendo per dare risposte ai bisogni immediati dei cittadini possa essere ripagato con una maggiore crescita. Le due chiavi che Italia Viva da tempo sostiene essere necessarie per poter portare il Paese ad una crescita stabile e sostenibile sono quelle della riforma dell'Irpef dell'Irpef e dell'uso strategico delle risorse del *recovery plan*; quindi un uso di risorse distribuito non su tanti progetti vecchi nei cassetti, ma su un'idea di sviluppo del Paese che sia frutto di una visione che permetta di avere una grande riforma industriale della nostra Nazione. Le risorse di questo scostamento serviranno - così come il Governo ha indicato - per nuovi interventi a tutela del lavoro, per il sistema dei trasporti pubblici e per le Forze dell'ordine. Stanziamenti aggiuntivi sono previsti per il settore sanitario, anche in relazione alle necessità legate all'acquisto, alla conservazione logistica dei vaccini e dei farmaci anti-Covid.

con ristori anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, prestando attenzione a quei settori - quello del turismo, quello montano, soprattutto con riguardo al turismo invernale - che risultano essere enormemente schiacciati in questa crisi. Appare inoltre evidente che saremo chiamati a gestire un'importante campagna vaccinale, dovendo ancora una volta far fronte agli aspetti straordinari ed emergenziali legati alla pandemia. avevamo più volte sottolineato la necessità di aprire una discussione seria in quest'Aula non solo sul *recovery fund*, ma in generale sul futuro del nostro Paese; una discussione franca e non ideologica anche su uno strumento come il che ci avrebbe permesso di poter contare su più risorse per il nostro Sistema sanitario, pagando peraltro meno interessi e che avrebbe liberato ulteriori risorse per altri comparti, al fine di sostenere imprese e famiglie.

che ci possa essere una possibilità per superare la crisi che stiamo vivendo, che la si voglia affrontare e si voglia aprire una discussione seria e reale, magari anche aspra, che tenga conto del rispetto delle posizioni di ognuno e della necessità di fare sintesi su una posizione comune. Dalla relazione si evince che il Governo ha inoltre previsto che una parte dei 32 miliardi che ci apprestiamo a reperire con questo scostamento saranno utilizzati per il sostegno ai livelli di governo decentrati e al sistema delle autonomie. Ecco, sul punto io penso che dovremo lavorare affinché nei prossimi mesi si riesca a mettere i livelli istituzionali più prossimi ai cittadini nella condizione di rispondere alle esigenze di questi ultimi. con lo sblocco dei licenziamenti e con l'acuirsi delle difficoltà commerciali, degli artigiani e dei lavoratori autonomi, le sofferenze e la crisi sociale si manifesteranno nelle nostre città in modo più netto e crudo. Penso anche a cosa produrrà

Lo dico in modo chiaro: facciamo in modo che quelle istituzioni siano messe in grado di far fronte alle difficoltà che arriveranno. Non lasciamoli soli, diamo loro la possibilità di dare risposte concrete anche a quei bisogni.

Aggiungiamo e sommiamo altri 32 miliardi di debito pubblico che pagheranno le future generazioni, che avranno come ipoteca sul proprio futuro 132 miliardi di euro; i primi 100 approvati fino al mese scorso e i 32 che approviamo oggi - attraverso l'autorizzazione che certamente Camera e Senato daranno - che si vanno ad aggiungere ai 40 miliardi che abbiamo appena approvato attraverso la legge di bilancio del dicembre 2020. Purtroppo i precedenti non depongono a favore del Governo, oggi, in quest'Aula, praticamente assente

ma solo una maggioranza relativa, che non è stata altro che un'accozzaglia di parlamentari, i quali certamente vi presenteranno il conto quando ci saranno da spendere i 32 miliardi. Una domanda è perciò d'obbligo in questo momento: con quale serenità e con quale spirito d'animo oggi noi siamo qui a votare il nuovo scostamento? C'è una sola parola: responsabilità.

Il vostro modo di spendere le risorse degli italiani si è dimostrato fallace, ha fatto acqua in tutti questi mesi e noi non vogliamo proseguire e andare oltre,

per tutte le attività che avete chiuso per decreto in questo ultimo anno. Oggi abbiamo il ministro Gualtieri, nell'audizione che abbiamo svolto in Commissione bilancio, ha ha confermato che occorre un cambio di passo anche per quanto riguarda queste somme da risarcire ai contribuenti italiani; tuttavia gli abbiamo detto che ormai il tempo è scaduto perché dopo questo ulteriore scostamento ci ha chiaramente detto che non ce ne saranno altri. ce ne saranno altri. Ci tengo poi a sottolineare l'incoerenza di fondo che avete perché mentre oggi ci chiedete di autorizzare un ulteriore scostamento di 32 miliardi, tra due settimane, cioè non più tardi del 31 gennaio, gennaio, l'Agenzia delle entrate ripartirà con oltre 30 milioni di cartelle esattoriali, quindi con una mano date e con l'altra prendete e togliete queste briciole che oggi stiamo dando ai contribuenti italiani.

Noi invece pensiamo che ogni impresa meriti di vivere di luce propria, soprattutto se ad affossare queste imprese sono state le vostre decisioni scellerate. Avete cercato responsabili e untori ovunque, nelle palestre, nei ristoranti, nei bar, nei cinema, sulle piste da sci; eppure, dati alla mano, la nostra Nazione purtroppo

mancette, prebende e quindi qualche migliaio di euro in prestito a fondo perduto che farete vivere le tante attività che in questo ultimo anno avete ridotto allo stremo. Conoscete le proposte che abbiamo fatto. Il nostro *leader* Giorgia Meloni ha detto in mille modi che bisognava cambiare percorso, strada e atteggiamento, ma voi chiaramente siete sempre stati sordi nell'ascoltare le nostre proposte che desidero ricordare. Abbiamo detto che i ristori non vanno assegnati in base ai codici Ateco, ma in base al calo di fatturato,

e non continuare a stare attaccati alle vostre poltrone, perché i veri responsabili siamo noi di Fratelli d'Italia, che da mesi, dentro e fuori questo Parlamento, facciamo proposte che questo Governo non ha mai voluto ascoltare.

Dopo la giornata di ieri, che non ho avuto difficoltà a definire artificiale, abbiamo questa giornata che ha invece più a che fare con il futuro dell'Italia

impegnare le risorse che ci saranno nel futuro guardando al passato, oppure guardando al tempo nel quale, poi, le opportunità riguarderanno le giovani generazioni. Noi ci stiamo occupando di fare in modo che l'Italia ritrovi la via del futuro, facendo sì che le migliaia di attività nei diversi settori del lavoro e dell'economia trovino copertura, trovino copertura, strumenti e possibilità di riscommettere con fiducia nei confronti di ciò che è stata la fonte del loro reddito. Pensate ai bar, ai ristoranti, alle attività alberghiere e a quegli interstizi di attività digitali che sono a supporto della nostra collocazione turistica nazionale e internazionale.

la classificazione, che collocava in rubrica le attività per come sono state conosciute dai Ministeri vigilanti e da quelli che hanno avuto a che fare con la promozione economica. Adesso arriva il turno di sostenere quelle attività che non hanno la rubrica dei codici Ateco, ossia le filiere, che sono poi la verità dell'economia.

attività. Se il bilancio dello Stato non presentasse possibilità di flessibilità davanti alle rotture di civiltà e alle interruzioni a valenza ciclica dell'economia, noi avremmo un bilancio feticcio, un bilancio totem. Per fortuna il bilancio ha la possibilità di compiegarsi rispetto alla crisi, recuperando margini di mobilità, flessibilità e compiegamento che consentiranno ai singoli settori di attività di ricominciare. Questo vale anche nel rapporto con il quadro comunitario di sostegno: 32 miliardi di euro verranno infatti collocati nel circuito dell'economia reale. Qual è il compito del Parlamento? Non organizzare la politichetta del conflitto, che organizza la visibilità a tutti i costi, di Narciso, dell'estetica del dire della ricerca dell'estetica dell'esserci. Serve invece monitorare e fare in modo che tutti gli elementi della realtà pervengano alla normazione normazione e che nessuno sia escluso, perché in queste prime fasi abbiamo avuto involontariamente dei settori segnati da esclusione. Le lamentele dei settori minori dell'artigianato e del commercio e di quegli interstizi della collocazione turistica e delle agenzie di viaggio ci danno carichi di lavoro.

valorizzando l'interoperabilità dei dati di cui Sogei dispone. Non è possibile che nel 2021 ragioniamo ancora senza valorizzare il patrimonio conoscitivo di cui disponiamo. Cito un fatto. Ai tempi del Giubileo ad alta densità partecipata che impegnò tutti i livelli dell'ordinamento, nel 2000, si riuscì, con i dati che avevamo, a sapere esattamente chi sarebbe arrivato a Roma quel giorno, con quale livello di devianza - diciamo così - valutabile in anticipo. Quindi i dati ci sono per far sì che la macchina della normazione si adatti perfettamente alla realtà dell'economia. Su questo, noi dobbiamo osare di più, pretendere di più, compiegare, organizzare flessibilità, facendo in modo che tutta la realtà entri nella norma, tutta la realtà economica trovi copertura, supporto e sostegno. Bene la misura riguardante, per esempio, le autonomie locali, misura derivante dai 32 miliardi di euro. Bene le risorse riferite alla riuscita della vaccinazione. Il vaccino è compito della comunità scientifica; la vaccinazione è compito dell'ordinamento istituzionale e dell'ordinamento delle autonomie sanitarie territoriali. Dobbiamo fare in modo che la vaccinazione significhi vaccinatori in numero sufficiente; dobbiamo fare in modo che scatti anche una dimensione culturale di convincimento: vaccinarsi

di ciascuno. Le misure sono significative, anche quelle riferite al *recovery plan*, perché esso contiene misure che aiuteranno i territori a ripartire sul piano della modernizzazione, della transizione energetica digitale, della transizione verso un futuro che porterà più diritti e opportunità. Che fa la politica su questo? Fa da spettatrice o organizza monitoraggio, indirizzo, riordino e recupero di risorse non spese, con una nuova graduatoria di priorità in ragione di ciò che di volta in volta la realtà ci imporrà? Noi dobbiamo tenere a bada, però, il feticcio della lotta politica a tutti i costi, anche quando l'ordinamento richiederebbe univocità, unità e senso di responsabilità. Ma come si fa, in un momento nel quale nazionale ed internazionale corrispondono, per la qualità della paura, della preoccupazione e del timore, a far sì che si divida uno Stato nazione, che si divida una comunità di classe dirigente, avendo l'urgenza dei problemi, la disponibilità delle risorse e l'aspettativa della cittadinanza che le decisioni accadano. Su questo ieri non è stato all'altezza il dibattito complessivo del Parlamento. Noi dobbiamo fare in modo di recuperare le ragioni delle urgenze e le ragioni del ruolo di ciascuno. Naturalmente, il mio è un contributo affinché votino tutti a favore dello e ci costituiamo come una comunità che indirizzi e porti più realtà possibile dentro ai luoghi della decisione. Signor Presidente, ho dato il

Grazie

perché oggi, francamente, votare questo scostamento sul piano politico è imbarazzante.

che era giusto che mi facessi "violentare" nell'interesse esclusivo delle imprese e delle famiglie. Cari amici, ho fatto due conti: in

presenti in Aula. Oggi stiamo parlando di uno scostamento da 32 miliardi di euro e non siete neanche in Aula. *(Applausi)*. E meno male che è arrivato il vice ministro Misiani. Il Governo è assente, mentre quando si tratta di salvaguardare la posizione, tutti presenti uno dopo l'altro; anzi, portiamo anche qualcuno col Covid! Ci avete provato, ma non vi è riuscito ieri, però ci avete provato. Oggi che si parla dell'interesse reale della Nazione - 32 miliardi di euro che spenderete male, come al solito, come avete fatto con gli altri 120 miliardi che avete fulminato in nove mesi di assoluta, totale incapacità di Governo - non c'è nessuno. *(Applausi)*. Io lo so perché non ci siete: perché avete vergogna di dire che ci spillate altri 32 miliardi che saranno uno zaino negativo sulle spalle delle future generazioni. Eppure, non paghi di questo, continuate a darvele di santa ragione. Grazie al collega Dal Mas, che è uomo attento, sono andato a recuperare l'intervento del collega Primo Di Nicola che, riferendosi alla senatrice Bellanova - ricordando Macaluso - l'ha definita l'ha definita politico di seconda fila che, per lucrare posizioni di potere non meritate, sfrutta la qualifica di bracciante. Ebbene, vi dovete vergognare anche di quello che pensate, non soltanto di quello che dite. E giù, botte secche tutti i giorni. Ieri, francamente, durante il dibattito - non mi nascondo - ho mandato un messaggino WhatsApp al capo di Italia Viva e gli ho scritto: «Ma dopo tutto quello che ti hanno detto oggi in Aula tu ti astieni?

Quindi, mi sono fatto convincere e voterò a favore dello scostamento; ma lo facciamo, come Forza Italia, soltanto nell'interesse delle famiglie e delle imprese e vigileremo attentamente come spenderete e investirete questi soldi. Per il momento, fossi in voi, mi vergognerei. Per il resto, ci penseremo più avanti.

siamo già al primo scostamento; non uno scostamento da poco, ma uno scostamento che è un'altra legge di bilancio: 32 miliardi. Sono 32 miliardi di cui l'economia italiana ha bisogno, ma verranno davvero utilizzati per dare impulso e aiuto al tessuto produttivo e sociale del nostro Paese? Paese? Mi auguro che questo nuovo indebitamento vada veramente a beneficio della nostra economia. Le breve descrizione degli intenti del Governo, contenuta nella relazione, prevede nuovi stanziamenti a tutela del lavoro - e va bene - la cassa integrazione, sostegno alle autonomie locali e risorse per la Protezione civile e le Forze dell'ordine, per il settore sanitario e per i trasporti pubblici. Purtroppo, solo in fondo alla lista troviamo la rimodulazione temporale dell'invio delle cartelle esattoriali, una delle battaglie a cui teniamo e, solo come ultimo punto, si citano una serie di misure in favore

Stiamo assistendo alla distruzione del tessuto sociale delle piccole e medie attività commerciali,

Gli operatori del turismo, della ristorazione, dello sport e della montagna chiedono di essere ascoltati. Hanno soluzioni, hanno adeguato le loro strutture alla richiesta di sicurezza dettata dalla crisi sanitaria non vogliono neanche i ristori, che soprattutto per le attività di medie e grandi dimensioni saranno sempre inadeguati, ma chiedono di poter lavorare in sicurezza.

per un fisco più semplice.» *(Applausi)*. Ascoltate la rabbia e lo sconforto degli operatori economici e cominciate ad ammettere anche gli errori

Viviamo qua dentro, ma fuori di qui il mondo reale sta attraversando una crisi senza precedenti. Ho molti dubbi sul reale utilizzo di questi 32 miliardi di euro. In Commissione bilancio abbiamo chiesto una stima di come verranno suddivisi questi denari, il vice ministro Misiani mi ha risposto francamente e voglio che sia messo agli atti anche in questa sede. Il Vice Ministro ci ha fornito una stima, pari a due terzi dell'intero importo, che andrà in favore del tessuto economico e delle imprese.

inizio il mio intervento con un ringraziamento per tutti quelli che, con alto senso delle istituzioni, della giustizia e considerazione per il futuro del Paese, hanno inteso votare nella giornata di ieri per continuare un percorso del quale la votazione di oggi è solo un ulteriore importante passaggio. Vivere in continua contraddizione con la propria ragione è moralmente intollerabile. La strategia spinta, il sotterfugio, lo stratagemma spesso e volentieri sono solamente la via più semplice verso la schiavitù della libertà. Siamo al paradosso che oggi per alcuni colleghi sembrerà del tutto normale votare l'ennesimo scostamento di bilancio, così come hanno votato la proroga dell'emergenza, quando, allo stesso tempo, hanno posto dei distinguo sul *recovery fund* e addirittura avallato il ritiro di due ministri dal Governo sulla base di discorsi pretestuosi. Mentre qualcuno antepone la propria carica al bene comune, noi abbiamo confermato senza indugio la fiducia a questo Governo, capace di attuare politiche emergenziali e al contempo di mettere in campo misure di più ampio respiro, che promuovono un'idea di società basata sulla giustizia sociale e sull'inclusione. Tante sono le sfide che abbiamo vinto, tante quelle che ci attendono quando usciremo da questa crisi e dovremo ripensare la nostra quotidianità e immaginare un nuovo modello di socialità. crisi attuale non è solo sanitaria; è una crisi sociale ed economica, ma è anche una grande opportunità per riflettere sul nostro sistema e le nostre relazioni. Il nostro futuro dipende da quali strumenti sapremo mettere in campo per chi si è trovato in ginocchio a causa della mancanza di lavoro, per la perdita dei cari o per il venir meno di quel tessuto sociale alla cui protezione non abbiamo per un solo momento cessato di lavorare. Noi ne siamo consapevoli; chi ha sospeso il proprio appoggio al Governo non credo. Se a voi questo sembra normale, a me no e nemmeno agli italiani. Ma se poi andiamo nel dettaglio a vedere chi ha votato positivamente tutti i precedenti scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento, vediamo come anche tutti voi che siete seduti tra i banchi dell'opposizione, siete stati concordi sulla necessità di proteggere l'economia italiana e le aziende in crisi, fornendo supporto economico a questo piano. Quindi come funziona? Senatore Mallegni, la responsabilità è a corrente alternata? Quando pochi secondi fa parlavo di un atteggiamento al limite del lunatico, quasi votato alla schizofrenia, da parte di un ex *partner* di Governo, posso sicuramente allargare questo ragionamento anche all'opposizione. Che senso ha oggi essere concordi sulla necessità di ulteriori 32 miliardi per supportare i tanti settori in difficoltà, quando poi, se dovete votare una legge di bilancio, negate puntualmente la fiducia al Governo da cui non vi sentite rappresentati? rappresentati? Anche la legge di bilancio faceva parte del piano di ripresa. Sono certo che siamo tutti concordi, in quest'Aula, sulla necessità di stanziare quante più risorse possibili. Una fase come quella contingente però vorrebbe unità nel lavoro di tutti i giorni. Attenzione però: bisogna smettere di provare ad ogni passo lo sgambetto a questo Governo. Chi evoca l'arrivo di un Governo cosiddetto nazionale lo fa solo per il proprio tornaconto, non certamente per il bene degli italiani. Tutto ciò è opera di chi ha aperto una dissennata crisi, voluta non già da quello che veniva definito il Telemaco rottamatore, che torna ad Itaca a caccia degli usurpatori dell'isola; chi ha cercato di riportarci alle urne, in realtà, ha cercato di usurpare un ruolo, quello del presidente Conte, che ha dimostrato il proprio rigore ignorando ricatti e lusinghe. Oggi il Governo chiede l'autorizzazione a uno scostamento di ulteriori 32 miliardi, oltre i cinque scostamenti già autorizzati lo scorso anno: sei grandi interventi per raggiungere le risorse necessarie a fronteggiare la crisi. Nessuno deve essere lasciato indietro e quindi, se necessario, potremo valutare ulteriori scostamenti anche in futuro. in futuro. Spero veramente però, che con la primavera e con l'avanzamento del piano vaccinale, la pandemia si possa sconfiggere e si possa ritornare ad una normalità per tutti i settori economici e produttivi. Tornando al tema di oggi, devo sottolineare come il MoVimento 5 Stelle sia sempre stato in prima linea per fornire il maggior supporto possibile a tutte le categorie: i miliardi di oggi serviranno per rifinanziare la cassa integrazione per i prossimi mesi; saranno ossigeno fondamentale per tutto il settore Horeca (Hotel, ristoranti, bar), per il comparto del turismo invernale, per il settore dell'intrattenimento, per i cinema e per i teatri, insomma per tutti i colori a cui stiamo chiedendo ancora degli importanti sacrifici. Ovviamente di questi miliardi beneficerà anche la scuola, una scuola finalmente tornata in presenza (era ora), anche se non con orario pieno, ma questo rappresenta l'emblema del ritorno ad una parziale normalità. Il lavoro di questo Parlamento non finisce con l'approvazione dello scostamento odierno ed occorre velocemente stabilizzare la maggioranza. Conte ha ed avrà la nostra fiducia, perché non ha anteposto il suo ego al bene del Paese. Il governo Conte ha azzerato le individualità, bandito i protagonismi, creato una squadra coesa che ha avuto come unico e solo obiettivo farci uscire da questa crisi sanitaria, economica e sociale. Chi, invece, questo senso dello Stato non ce l'ha, forse perché offuscato da mire personali mai sopite, vive del conflitto e chiude le porte alle grida di aiuto della gente. Il voto di ieri ha dimostrato che anche nel Gruppo che voleva la crisi ha fatto breccia il principio di realtà. Fortunatamente non tutti sono pronti a gettare l'Italia al vento. Chi ha voluto la crisi vada come Icaro verso il suo sole e disgiunga finalmente la sua china da quella della Nazione. Noi andiamo avanti senza timore e, come dice spesso mia madre, male non fare, paura non avere.

Signor Presidente, solo alcuni minuti per ricordare gli interventi che sono stati fatti e le proposte che sono state avanzate, sia dalla maggioranza che dall'opposizione, sull'utilizzo di queste risorse e magari anche di altre che sarà necessario mettere in campo per dare risposte concrete a chi oggi purtroppo non può lavorare per via delle restrizioni e per la crisi pandemica. Vorrei quindi ringraziare veramente tutti coloro che sono intervenuti, sia della maggioranza che dell'opposizione. La

che servono ai cittadini e alle aziende, che hanno bisogno. Sarà quindi un modo poco razionale, sembrano soldi gettati al vento, ma in realtà sono indirizzati alle persone che hanno veramente bisogno.

che sia un'idea che il Governo porta avanti, cui darà veramente concretezza. Il collega D'Alfonso ci ha ricordato che bisogna efficientare la pubblica amministrazione e sono d'accordo, anche perché, con le risorse del *recovery* *fund*, si farà il possibile per riuscire a migliorare ogni procedura e ogni processo amministrativo. La senatrice Corrado ci ricordava di tutelare il

non stanno spendendo. Dobbiamo ricordarlo ed è una cosa molto delicata da affrontare, perché spesso si può andare incontro a critiche. Ci è stato anche consigliato di fare in modo che le risorse vengano utilizzate nel modo migliore possibile per incentivare e incrementare il *business*, le attività delle imprese, il lavoro.

ma anche dalle imprese. Infatti, se guardiamo ai dati della Banca d'Italia, ci accorgiamo che ci sono più di 140 miliardi di euro di nuovo risparmio. Secondo me dovremmo veramente concentrarci, tutti insieme, e trovare la formula più adatta e più sicura per fare in modo che questo risparmio

Allo stesso tempo non si può non ricordare l'aumento del debito pubblico: siamo arrivati a 155 miliardi in più per gli stanziamenti, per i ristori e per i lavoratori. Non sono però somme che lo Stato ha speso per una mancata *spending review*, per inefficienza o inefficacia nei processi; no, sono soldi che abbiamo speso perché le famiglie hanno bisogno di andare avanti.

quindi al Governo e al Ministero dell'economia e delle finanze di fare il possibile affinché tale riflessione venga portata nelle sedi istituzionali europee e si trovi anche in questo caso una soluzione compatibile con le nostre esigenze per cercare di rendere gestibile e sostenibile il nostro debito pubblico, soprattutto per la parte riferita alla crisi pandemica. Detto ciò, circa

Signor Presidente, desidero ringraziare, a nome del Governo, i Gruppi di maggioranza e di opposizione, le senatrici e i senatori che sono intervenuti nel dibattito odierno. Li ringrazio ed esprimo l'apprezzamento per i contenuti e per i toni emersi nel dibattito. Lo scostamento che ci apprestiamo a votare, i 32 miliardi 32 miliardi per i quali il Governo ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione, rappresentano un atto importante. Non a caso, la Costituzione prescrive la maggioranza dei componenti, non la maggioranza semplice, per l'approvazione degli scostamenti di bilancio. Questi 32 miliardi rappresentano debito aggiuntivo che ricadrà sulle generazioni future del nostro Paese. Questo ci carica di una responsabilità importante e del dovere di utilizzare al meglio tali risorse per aiutare le famiglie, i lavoratori e le imprese del nostro Paese, che devono far fronte ad una situazione molto difficile di emergenza sanitaria, economica e sociale. Credo che il voto unanime del Senato nei confronti di questa richiesta possa essere un segnale molto importante, un segnale di unità e di lavoro comune e condiviso nell'interesse generale del Paese verso la comunità nazionale italiana. Sulla

Prendo atto di quanto ha detto il senatore Calderoli. di risoluzione, daremo la parola al senatore Faraone, che dovrà dirci quel che pensa in ordine a questo e quel che pensa il Governo.

e alla Presidenza viene presentata formalmente questa, devo considerare questa e non posso considerarne altre. La vuole mettere in distribuzione, perché anche noi possiamo sapere cosa votiamo?

al rappresentante del Governo di darmi un parere sulle tre proposte di risoluzione che ho in mano - e mi risultano, dal Segretario Generale, essere state distribuite esclusivamente queste tre, è evidente che non posso essere a conoscenza di una quarta, che non ho e che mi dicono non essere stata distribuita. Occorre che ci sia chiarezza fra di noi, perché non ho alcuna difficoltà a dire se questo è un testo 2. Presidente, a questo punto mi rendo conto

E, se è stata distribuita soltanto la seconda, questo significa che c'è corrispondenza fra quello che è dato alla Presidenza e quello che è stato distribuito ufficialmente e formalmente in Aula.

Credo sia politicamente importante che la risoluzione su cui il Governo esprime parere favorevole rifletta nei contenuti un confronto che va al di là del perimetro della maggioranza.

colleghe e colleghi, naturalmente il nostro Gruppo voterà a favore del nuovo scostamento di bilancio. Purtroppo pensiamo che questo non sarà l'ultimo e che nei prossimi mesi ci vorrà un ulteriore intervento, perché la pandemia non è per niente finita e, come ha sottolineato l'Ufficio parlamentare di bilancio, difficilmente ci sarà il rimbalzo del 6 per cento immaginato la scorsa estate. Spero di sbagliarmi, perché è davvero pesante l'eredità che rischiamo di lasciare sulle spalle delle prossime generazioni. Per questo, dobbiamo spendere con grande cura tali risorse per aiutare i lavoratori e le imprese ad affrontare l'attuale difficilissimo passaggio

Si deve superare innanzitutto il criterio dei codici Ateco con quello delle perdite di fatturato, seguendo l'esempio degli altri Paesi europei. La base temporale di riferimento deve essere l'anno solare e non il semestre, perché solo così non lasceremo fuori le aziende e i lavoratori stagionali. In particolare, come annunciato dal ministro Boccia, il prossimo decreto-legge ristori deve avere in cima alle priorità i lavoratori e le imprese di montagna, che sono stati i più duramente colpiti dagli ultimi DPCM, poiché la stagione invernale non è neppure potuta iniziare.

Bisogna non solo prorogare quegli adempimenti fiscali la cui scadenza è prevista per il prossimo 31 gennaio, ma occorre anche avviare il percorso per una nuova pace fiscale, con una serie di interventi che prevedano per le categorie più drammaticamente colpite un vero e proprio anno bianco fiscale e la possibilità di un nuovo saldo e stralcio, a cominciare dai contenziosi di piccolo importo. Serve un occhio di riguardo per i liberi professionisti. Con l'ultimo decreto ristori e con la legge di bilancio sono state introdotte misure in un certo senso storiche, come gli ammortizzatori sociali per una categoria di lavoratori che ne era completamente sprovvista. Lo sforzo che bisogna fare in questa fase è sempre quello di trovare un punto di equilibrio tra aiuti e strumenti che incentivano la ripartenza. sulle partite IVA si potrebbero rivedere i criteri per l'accesso e la durata del regime dei minimi, nonché quelli per aderire al regime forfettario. Occorre soprattutto un deciso investimento su tutti gli strumenti che sono in grado di fare da moltiplicatore economico. Se n'è discusso diffusamente in questi giorni, quindi mi limito solo a una riflessione: alla fine di quest'anno il rapporto tra debito e PIL andrà oltre il 160 al periodo precedente alla pandemia. Non possiamo immaginare di sostenerlo con i *trend* di crescita che l'Italia ha conosciuto negli ultimi vent'anni e che l'hanno vista fanalino di coda in Occidente. Per questo occorre gettare le basi per un Paese che, superata l'emergenza e la stagione degli aiuti europei, sia in grado di crescere ai livelli del resto d'Europa. Quello che voglio dire è che l'Italia più di tutti ha bisogno di un *recovery plan* come strumento per la modernizzazione e per la competitività del proprio tessuto produttivo. Non è una partita importante; è una vera e propria partita della vita. Non è però solo ai progetti del *recovery* che dobbiamo guardare. Una dinamica economica positiva può essere favorita anche da semplici riforme che non richiedano ingenti investimenti economici. Penso, come sempre, alla semplificazione burocratica e di quelle procedure che, mai come in questi mesi, hanno dimostrato quanto rappresentino un ostacolo e un problema. Senza una profonda rivisitazione del codice degli appalti, ad esempio, non saremo mai in grado di attuare i progetti del *recovery*, perdendo risorse che sono la nostra occasione per rilanciare il sistema. Penso alla riforma della giustizia, ma anche a tutti gli altri interventi che andremo a scrivere in quest'anno. Ogni aiuto non può essere fine a se stesso, ma deve indicare una prospettiva di ripartenza, perché non bisogna solo resistere, bisogna tornare a esistere e a creare sviluppo. Per concludere, signor Presidente, sono davvero grandi lo sforzo e l'impegno che ci aspettano; sono davvero tante e tutte importanti le questioni di cui dobbiamo occuparci. È questa la ragione per la quale ieri abbiamo votato contro una crisi di Governo che oggi il Paese non può assolutamente permettersi. Il tempo, mai come oggi, non è una variabile secondaria: basta pensare semplicemente alle scadenze di fine gennaio. Se questa crisi continuerà, rischiamo di fare tardi su una serie di questioni - e qui c'è tutta la partita sul *recovery* - perché c'è la situazione della diffusione del virus che va guardata con grande attenzione, vista la campagna vaccinale su cui neanche un solo minuto può essere perso. Questa è l'ora del massimo impegno, in cui serve una maggioranza forte e stabile, da costruire riscoprendo le ragioni del dialogo con chi c'è stato e trovando strade anche con chi da sempre si riconosce nei valori dell'Europa unita e solidale, con il confronto e il senso di responsabilità da parte di tutti. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) allo scostamento di bilancio.

Signor Presidente, stiamo discutendo oggi la relazione con la quale l'Esecutivo chiede al Parlamento l'autorizzazione ad aggiornare gli obiettivi di finanza pubblica.

ma anche a confermare una vocazione europeista, perché questo scostamento avviene grazie a un quadro regolatorio europeo che ci permette, da ormai un anno, di attuare scostamenti e di lavorare verso una politica espansiva che possa sostenere il tessuto economico e tutte le misure sociali e sanitarie. Con questo spirito, quindi, ci apprestiamo di bilancio per ulteriori 32 miliardi a valere sul 2021. È il sesto scostamento che votiamo da quando è iniziato il periodo pandemico, che porta l'indebitamento netto aggiuntivo a 140 miliardi, dei quali sentiamo il peso

situazione del quadro economico e di finanza pubblica; è molto pesante per noi che lo stiamo approvando e lo sarà ancora di più per chi arriverà dopo di noi. Anche l'onere sul debito aggiuntivo e purtroppo su quello pregresso è molto importante. È vero che è temperato dalla politica monetaria della Banca

porre grande attenzione all'attendibilità del rientro rispetto all'obiettivo di medio termine. è particolarmente importante che ci concentriamo sulla crescita e sul PIL. Se è vero che in questo momento tutta la politica economica è strettamente legata con effetti uguali e contrari all'atteggiamento che che si è deciso di adottare privilegiando la salute e la salvaguardia degli individui, è vero anche che questo ci dice che abbiamo un'unica strada da perseguire affinché il nostro PIL e la nostra crescita possano tornare a essere tali da sostenere l'enorme debito che ci siamo accollati per aiutare l'Italia. Questa unica via è il piano vaccinale. So che non è una politica economica, ma è ad essa strettamente connessa. La responsabilità che ci investe di fare bene e di fare subito, di fare bene nell'approvvigionamento e nelle somministrazioni e di fare tutto il possibile affinché l'approvvigionamento sia tempestivo e velocissimo è strettamente connessa alla nostra capacità di uscire economicamente da quello che altrimenti può diventare solo che un *loop* in negativo. Anche questi ulteriori 32 miliardi devono essere letti in tale ottica. Dobbiamo utilizzare le risorse aggiuntive per sostenere

sul *deficit*. In questo senso è molto opportuno, dopo un anno di misure, riuscire a fare anche una valutazione di impatto su quelle che hanno funzionato e su quelle più efficaci, adottando anche un'ottica selettiva e cercando di capire all'interno dei singoli comparti quali imprese e quali individui devono essere aiutati e quali invece possono ricominciare a camminare sulle proprie gambe. Questo è infatti l'obiettivo finale.

ci stanno segnalando che sono particolarmente burocratiche e quindi, anche nell'ottica *recovery*, questa è un'indicazione. Occorre ristorare i settori chiusi che non sono ancora stati ristorati: il settore neve, quello della montagna, ancora una volta quello turistico e quello crocieristico, che non ha potuto lavorare in tutto il periodo invernale. Bisogna introdurre la clausola perequativa, chiaramente per ristorare in maniera equa

misure attive sul lavoro. Se c'è una cosa che possiamo fare, mentre i nostri lavoratori sono obbligatoriamente fermi, è fare in modo di riqualificare le loro competenze in chiave digitale e *green*, seguendo le nuove

da una giornata nella quale l'intera Assemblea del Senato ha fatto una pessima figura, non solo davanti al popolo italiano, ma a tutta quell'Europa che ci ha guardato certamente non perché eravamo sovranisti o meno, ma perché il mercimonio che ha caratterizzato certe fasi e certi momenti della giornata e delle ore di ieri è veramente una pagina nera nella storia della nostra Repubblica.

stanziale attraverso la legge proporzionale. Dopo aver visto e sentito queste cose, signor Presidente e signori del Governo, oggi dobbiamo - o dovremmo - dare l'assenso allo scostamento di bilancio. Ebbene, signor Presidente, lo faremo con il senso di responsabilità che abbiamo, non verso il Governo, e con quel concetto di responsabilità che non ha niente a che vedere con il concetto di responsabili o meglio di irresponsabili che ha caratterizzato la giornata dell'evitata crisi di Governo di ieri. Lo faremo per senso di responsabilità verso i lavoratori italiani, dipendenti e autonomi, verso le partite IVA e i professionisti colpiti dalla mala gestione del *lockdown* e dall'incapacità di garantire regole di sicurezza che avrebbero permesso a tutti di restare aperti e di lavorare. - appunto - di questi *lockdown*, oggi siamo costretti a indebitarci ulteriormente per garantire almeno un adeguato ristoro alle nostre partite IVA. Oggi siamo di fronte a una barriera che stiamo per andare a sfondare, quella dei 170-175 miliardi di indebitamento, che rappresentano un macigno enorme per i nostri figli, per i nostri eredi. Il peggio è che questa marea di miliardi, che mai avremmo pensato di dover utilizzare, non viene nemmeno minimamente investita in misure strutturali, ma di fatto perlopiù impiegata in *bonus* assistenziali. quindi di una situazione davvero pesante, per la quale però perlomeno siamo riusciti a ottenere qualche assicurazione dalla maggioranza rispetto al

ristori i contributi a fondo perduto arriveranno anche ai professionisti. Il Ministro si è impegnato oggi in audizione e lo aspettiamo al varco nelle prossime settimane. Siamo felici che - come sembra - tra le promesse ci sia il superamento dei codici Ateco, una logica che di fatto

accettiamo queste promesse, sperando che siano reali e che il riconoscimento dei costi fissi sia un altro paradigma che ispirerà il Governo nel nuovo decreto ristori-*quinquies*. concludere, utilizzando gli ultimi due minuti che dovrebbero spettarmi. Serve però un cambio di passo. Apprezzo quanto detto anche dalla collega Conzatti, di Italia Viva, che mi auguro abbia la forza di portare

è rimasta una capace solamente di guardare ai redditi di cittadinanza o ce n'è ancora una che si ricorda che gli investimenti pubblici, in certe fasi economiche e storiche, dovrebbero essere un punto di riferimento per la ripresa del Paese?

che venga presa in considerazione anche la moneta fiscale e che finalmente vengano discussi in Commissione finanze e tesoro i disegni di legge trasversali sui crediti di imposta e la circolarizzazione della moneta per avere un mezzo che dia più risorse ai nostri cittadini.

una misura straordinaria, perché la fase che vive il Paese è straordinaria, a causa della pandemia in corso, che ci costringe a prendere misure straordinarie per limitare i danni economici e sociali che stanno mettendo in ginocchio il nostro Paese. Questo ulteriore scostamento si è reso necessario perché l'evoluzione dell'epidemia, nella seconda ondata del virus che in tutto il mondo era stata prevista, ma che non si è riusciti a evitare nella sua recrudescenza e diffusione, sta colpendo la nostra economia in maniera ancora più drammatica rispetto ai primi mesi della scorsa primavera, perché infierisce su un corpo già ampiamente debilitato. E anche se le misure che sono state prese sino a oggi hanno permesso di evitare una chiusura totale del Paese, come nella prima ondata della pandemia, per contemperare l'esigenza di minimizzare i costi economici con quella di fronteggiare l'emergenza sanitaria, ciò non riesce a limitare più di tanto un effetto potenzialmente devastante sul tessuto economico, con un aumento esplosivo della povertà e delle diseguaglianze, non solo nelle aree più periferiche e degradate del Paese. il Governo ha affrontato le conseguenze economiche delle misure sanitarie adottate a partire dalla fine di ottobre attraverso l'adozione di quattro decreti-legge (i cosiddetti decreti aventi prevalentemente effetto per l'anno 2020, e delle misure recate dalla legge di bilancio 2021. Tuttavia, le principali stime economiche descrivono un peggioramento della congiuntura nello scorcio finale scorcio finale dello scorso anno, con un quadro economico aggiornato in cui, dopo un rimbalzo del terzo trimestre del tasso di crescita del PIL reale rispetto al trimestre precedente si è verificata una contrazione, nel quarto trimestre del 2020, che porterebbe la contrazione annuale in linea con la stima presentata nella Nota di aggiornamento del DEF (meno 9 Questo scostamento servirà pertanto a contrastare nuovamente l'emergenza. Riguarderà il solo 2021, con un'autorizzazione pari a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto. Le stringenti misure sanitarie richiedono infatti di essere accompagnate da nuovi interventi di sostegno e ristoro di entità nettamente maggiore rispetto a quanto preventivato nella legge di bilancio 2021. Sarà quindi fondamentale il decreto ristori cinque, che nel giro di qualche giorno arriverà in Aula, per il sostegno ai settori più esposti alla crisi determinata dal Covid-19. Sarà importante che il provvedimento contenga misure a tutela dei lavoratori, compresa la possibilità di prolungare ulteriormente il blocco dei licenziamenti per non rischiare una drammatica crisi sociale. Sappiamo bene che l'epidemia potrà essere debellata quando verrà effettuata su ampia scala la somministrazione di vaccini efficaci, che rappresentano oggettivamente l'arma più forte contro il virus per il suo definitivo contenimento nei tempi più brevi possibili. Occorrerà certamente tempo perché la copertura vaccinale In Italia, il piano strategico per la vaccinazione stima che, nel quarto trimestre, si possa raggiungere una percentuale di popolazione vaccinata dell'ordine del 90 Siamo solo all'inizio. Dobbiamo fare in modo che questo tempo sia impiegato bene, con una puntuale organizzazione sul territorio. Dobbiamo approfondire meglio, perché, dopo un momento in cui l'Italia è stata prima in Europa per numero di somministrazioni di vaccino, da diversi giorni ci sono stati alcuni ritardi dell'azienda Pfizer nelle consegne e riduzioni nel numero di dosi, come del resto anche in altri Paesi europei. Dobbiamo adottare quindi interventi conseguenti, per non alterare il piano vaccinale nazionale. C'è ancora tantissimo da fare e dobbiamo correre molto velocemente per garantire il pieno successo di questa campagna. Ho pertanto trovato la posizione politica espressa nei giorni scorsi dalla vice presidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, inquietante, radicalmente sbagliata e culturalmente pericolosa. Ha fatto bene il ministro della salute Roberto Speranza a ribadire che il Servizio sanitario nazionale, tanto più in una grave emergenza sanitaria, ha l'obbligo di tutelare innanzitutto il diritto alla salute, a partire dai più deboli, da quelli che corrono più rischi di perdere la vita, indipendentemente dalla ricchezza dei territori in cui vivono. Colleghe e colleghi, la salute è un bene pubblico fondamentale. Il diritto alla salute è di tutti e non è un privilegio di chi ha di più. Il Paese ha davanti una sfida epocale. Le comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta di ieri in quest'Aula hanno avuto il merito di chiarire l'ampio respiro riformatore che servirà al nostro Paese per uscire da questa drammatica fase. Il *recovery fund* riveste un ruolo strategico nella ripartenza del nostro Paese, che necessita, in molti settori, di innovazioni e trasformazioni profonde, anche radicali, al fine di emergere da una condizione di crisi che da molto tempo ormai colpisce il nostro Paese. Ne discuteremo presto in Parlamento, apporteremo le nostre modifiche, se necessarie, e lo miglioreremo. È in gioco il nostro futuro. Nelle Commissioni bisognerà perciò lavorarci con rigore e serietà nell'esame complessivo credo sia giusto verificare e approfondire se gli investimenti per il Mezzogiorno siano adeguati per ridurre il divario accumulato con il resto del Paese ed effettivamente centrali nelle scelte politiche nazionali. Bene ha detto il presidente Conte quando ha sottolineato che un 50 per cento queste sono le stime - sarà destinato al Sud; altro che 34 per cento. L'Italia per ripartire ha bisogno della locomotiva del Sud: più ricchezza e più risorse per il Mezzogiorno perché, solo facendo correre il Sud, potranno correre il Nord e tutta l'Italia. Presidente, mi avvio alla conclusione con l'annuncio del voto favorevole allo scostamento di bilancio dei senatori di LeU e della maggioranza del Gruppo Misto. Ci rendiamo conto tutti della lunga e difficile giornata che abbiamo vissuto ieri con il voto di fiducia al Governo. La maggioranza è uscita più fragile, non c'è dubbio; per tutti comincia oggi una sfida, convinti di riuscire a rafforzare in Parlamento la maggioranza, per un patto di legislatura. Ora bisogna concentrarsi sui problemi degli italiani e lavorare intensamente; il Paese attende risposte rapide e noi dobbiamo essere all'altezza della speranza e della domanda di futuro dei cittadini: prima le persone.

valutazioni e interpretazioni dell'opposizione - desidero soffermarmi su alcuni aspetti che ritengo centrali, proprio perché oggi non stiamo compiendo un atto burocratico, ma una scelta politica di grandissimo rilievo. di grandissimo rilievo. Tutti i Gruppi parlamentari hanno richiesto al Governo di garantire la centralità del Parlamento anche nella gestione di una fase emergenziale; non possiamo partire dalla richiesta della centralità del Parlamento calpestando, ignorando o interpretando sul piano politico la Carta costituzionale. Non si garantiscono centralità e credibilità alle istituzioni piegando le regole della nostra democrazia. Lo dico con grande chiarezza: non possiamo confondere la maggioranza necessaria per garantire la fiducia a un Governo in carica con quella rafforzata necessaria per approvare lo scostamento di bilancio e le modifiche costituzionali. È una falsa caricatura politica, che offende la credibilità e la dignità di questo Parlamento. stiamo lavorando insieme - credo - il primo punto di partenza deve essere quello di riconoscere la scelta che oggi stiamo compiendo: 32 miliardi di indebitamento netto, 35 miliardi di fabbisogno, che è il saldo netto da finanziare, 40 miliardi in termini di competenza e 50 miliardi in termini di cassa. Sono nuovo debito, che inevitabilmente richiede un'assunzione di grande responsabilità. È evidente che la nostra Carta costituzionale, chiedendo una maggioranza rafforzata, indica la strada della condivisione e della responsabilità nazionale e considero positivo che in quest'Aula oggi, probabilmente, si raggiungerà un'unanimità necessaria, che rafforza la credibilità di questa istituzione.

dobbiamo considerare il senso delle parole che utilizziamo. Recuperiamo la credibilità delle istituzioni che rappresentiamo, proviamo a dare senso compiuto e profondità alle parole.

Smettiamo di usare termini incompiuti, privi di qualsiasi connessione con il senso etimologico delle parole. Il Ministro ha la funzione fondamentale di guidare il Paese fuori dalla pandemia dunque dobbiamo rappresentare la dignità di queste istituzioni, se vogliamo offrire ai cittadini la credibilità e la responsabilità nazionale, che in questo voto oggi si manifesta. Considero questo passaggio politicamente rilevante, perché significa che quando in gioco c'è il bene comune del Paese, la necessità di salvaguardare gli ammortizzatori sociali e di garantire alle imprese la liquidità necessaria per superare questa fase, l'ostinato lavoro teso ad accompagnare l'Italia fuori dalla crisi pandemica richiede giustamente il superamento degli steccati e delle barriere tra maggioranza e opposizione, mettendo in campo una condivisione necessaria, quando in gioco c'è il destino del Paese. Stiamo infatti parlando di questo ecco perché dobbiamo restituire credibilità e dignità alla politica. Lo si fa se, prima di tutto, tra noi riconosciamo la responsabilità delle Assemblee parlamentari e la credibilità dei provvedimenti che stiamo esaminando. Cominciamo a sfatare i luoghi comuni: dobbiamo riconoscere che non siamo all'interno di una fase economica, nella quale si possa parlare di ordinarietà. Chiedere ad un Governo di attraversare una pandemia, superando contemporaneamente nodi strutturali, economici, sociali e di disuguaglianza, che ci trasciniamo da vent'anni, non è degno della buona politica. La buona politica sa distinguere le fasi. stiamo portando l'Italia fuori dalla pandemia e sappiamo che dobbiamo unire, soprattutto col nuovo decreto ristori, la gestione emergenziale e una lettura compiuta della crisi pandemica, che inevitabilmente richiede una visione e risposte nuove, per creare crescita economica, per superare le disuguaglianze e per costruire un nuovo modello di sviluppo economico, con il nuovo volto dell'Europa. Questa è una sfida grande, enorme, che richiede responsabilità e sono orgoglioso che il Partito Democratico si collochi dalla parte della stessa, in questo passaggio così difficile e così delicato. È la nostra identità, sono le radici naturali della nostra appartenenza politica. Non dobbiamo avere paura nell'assumerci questa responsabilità e non dobbiamo neanche avere paura di chiedere, di sforzarci di allargare il confronto,

perché il distanziamento, che viene richiesto sul piano delle relazioni tra le persone, colpisce e rinchiude le giovani generazioni, chiedendo loro un sacrificio aggiuntivo, nella rinuncia ad una scuola in presenza, ma anche nella rinuncia a tante relazioni, che sono parte integrante della crescita e dello sviluppo delle giovani generazioni. allora che, con grande determinazione, dobbiamo riconoscere il lavoro che stiamo compiendo e agganciare alle misure emergenziali un progetto per uscire da questa crisi pandemica.

e crediamo che queste misure siano fondamentali, per non lasciare il mondo delle partite IVA nella solitudine e nell'indifferenza. Aver garantito l'universalità di un sostegno, che non c'era, è qualcosa di importante e prezioso, che deve andare oltre un dibattito assurdo sulle poltrone, sulle responsabilità e sulla fuga dalle responsabilità, che in questo momento credo non ci sia consentita. Non è consentito all'Italia scappare dalla responsabilità anche per le sfide europee che abbiamo di fronte, dove ci giochiamo il nostro futuro e il futuro dell'economia e della società italiana. Allora, Presidente, il nostro voto di fiducia oggi non è un voto burocratico, è l'interpretazione autentica della nostra identità, è uno stimolo per il Governo a superare il meccanismo dei codici Ateco e a cominciare ad interpretare le filiere come risposta adeguata per riconoscere i necessari sostegni, fondamentali per attraversare questa crisi, alle imprese che hanno perso fatturato, uscendo dal confronto mese su mese e da quei codici Ateco che probabilmente non sono in grado di interpretare per intero la filiera economica. economica. Credo che su queste operazioni, al pari della necessità di destinare nuove risorse per dare velocità al piano vaccinale*...

colleghe e colleghi, nella giornata di ieri il Governo ha ottenuto la fiducia da quest'Assemblea, ma non la maggioranza assoluta, pur essendo vero che i sondaggi vanno solo annusati e non presi per oro colato, sembra certo che non rappresenta la maggioranza degli italiani. Mentre voi consumavate i vostri intrighi, scontri o dibattiti di Palazzo per il Conte 2 in mutazione, fuori fuori un altro virus in mutazione, il Covid-19, ci ha fatto superare gli 80.000 morti e non si intravede ancora la fine. Un Paese ancora in completo disordine: Regioni multicolori, parametri che variano continuamente, senza un chiaro piano di vaccinazione e a oggi pare senza neanche la certezza di avere i vaccini. senza un quadro di regole, senza un piano per passare dai ristori almeno alla previsione degli accompagnamenti per la ripresa. È scarsa l'evidenza dei 150 miliardi finora spesi. Colleghi, a marzo 2020, il Covid-19 era uno spiacevole ed imprevisto evento. E passi l'euforia dei buoni vacanza, dei monopattini e dei rubinetti, ma da ottobre vi è coscienza di tre dati rilevanti: la seconda ondata

ferie forzate, come il primo *lockdown*, ma conseguenze di lungo periodo: chiusure, fallimenti, disoccupazione, sofferenza sociale. Ora è previsto uno scostamento di 32 miliardi di debito che si aggiungono agli oltre 50 già autorizzati e un impegno di competenza maggiore di 40 miliardi. Non si può prevedere solo ristoro o proroghe, anziché percorsi per uscirne, come per le cartelle esattoriali. È necessario un salto di qualità, un percorso di nuovo avvio per chi riesce ad avviarsi; regole anche temporanee che accompagnino chi purtroppo non riesce, imprese e lavoratori. quindi un intervento sul codice della crisi, interventi che riguardino Naspi, politiche attive del lavoro per chi è licenziato, perché arriverà questo momento. Quindi, l'azione non può essere solo assistenza temporale, peraltro minima purtroppo. Bisogna avere il coraggio di coniugare l'emergenza e la normalità.

lo scostamento odierno va in quella direzione), per il *recovery plan*, una sfida che vale tre volte il piano Marshall, stimabile in 90 miliardi per un percorso di regole di normalizzazione. Forza Italia ci sarà. Signori del Governo, signori della maggioranza che, come ho detto prima, non esiste totalmente, noi, manifestando la più sofferente preoccupazione sulla vostra capacità di finalizzare in modo efficace lo scostamento di bilancio che oggi ci viene richiesto, voteremo comunque a favore; a favore per l'Italia e per gli italiani, perché questo per noi è il senso di responsabilità.

ci riduciamo oggi, in poche ore, a votare lo scostamento di bilancio e non vedo, anche per il disinteresse generale, tutta questa apprensione. Stiamo facendo una cosa importantissima importantissima, lo ripeto - sulla quale, seppur in un brevissimo tempo, abbiamo cercato tutti di dare un contributo significativo.

ma soprattutto ha detto che bisogna essere efficienti, efficaci e selettivi. Ora, sul fatto che sia l'ultimo intervento (qualcuno l'ha già detto) forse c'è qualche dubbio, perché dipenderà da quanto sapremo essere precisi

aperture in sicurezza di tante realtà, a partire dalle scuole, dai trasporti e da tutte le attività che, tra l'altro, abbiamo dimenticato negli altri decreti Faccio un breve elenco, giusto perché abbiano almeno la citazione: i ristoranti, le palestre, i lavoratori dello spettacolo, della cultura, della musica, i teatri, i mercati all'aperto (una vitaccia per tutta la vita). Vorrei ricordare anche il blocco degli sfratti e la sofferenza dei piccoli proprietari immobiliari, che non sono dei miliardari riccastri, ma sono persone che, come tante altre, in un particolare momento storico, hanno pensato che l'investimento giusto fosse l'appartamento, la casa e che magari, con due o tre appartamenti e il blocco degli sfratti, si ritrovano in grandi ristrettezze. Ci sono tante ingiustizie da superare sicuramente.

del presidente Conte di ieri, le tante cose che non sono andate bene. Non saremmo seri se non lo facessimo. Allora serve ricordare quante cose non sono ancora

Lo Stato prima di tutto, evidentemente, perché certi passaggi li può fare solamente lo Stato attraverso il lavoro dei vari Ministeri.

non fare in modo che questa cifra così importante arrivi alle persone, ai cittadini e alle imprese. Il Gruppo Lega ha lavorato soprattutto perché ci fossero dei risultati importanti e ci fosse un ulteriore completamento per la decontribuzione delle partite IVA e degli autonomi;

più veloce, è però stato incredibilmente iniquo e sbagliato, perché riferito al mese di aprile su aprile, quindi non non corrispondente alla realtà delle imprese. Già questo superamento sarebbe un lavoro incredibile che permetterebbe di ristorare tante persone rimaste completamente escluse. Inoltre, il grande sforzo per il trasporto pubblico: una delle sfide più importanti per la sicurezza e per il contenimento del contagio è quella relativa al trasporto pubblico, sia per le attività normali

non possiamo ammazzare definitivamente con le cartelle esattoriali chi è già colpito dagli effetti del Covid sulla propria azienda e sulla propria attività. *(Applausi)*. Questa è un'altra cosa basilare

Dobbiamo pensare che questo futuro dovrà essere sviluppato e accresciuto da individui equilibrati, da ragazzi che possano avere uno sviluppo normale, equilibrato, senza particolari... Io non riesco ad ascoltare bene gli interventi e credo nessuno di voi, su un provvedimento così importante. Dicevo che abbiamo bisogno di individui equilibrati per affrontare gli effetti di questa pandemia, sotto il profilo economico e delle nuove povertà, ma anche per quanto riguarda il fatto di non poter uscire, di non poter avere una vita normale, un'attività fisica normale. Pensate a quanti

permettetemi di usare un'espressione gergale - stanno facendo uscire di testa troppa gente. E già si vedono, in modo più o meno

in un Paese dove ci saranno tante persone che avranno bisogno di assistenza, la cui efficienza non abbiamo ancora adesso.

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo, oggi il Parlamento è chiamato a pronunciarsi su un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi, per lo stanziamento di nuovi fondi volti a sostenere gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. Sono passati molti mesi dal primo scostamento di bilancio ed è impressionante pensare a quello che è accaduto in questo lasso di tempo, non solo in Italia, ma nel mondo. Siamo stati travolti da un qualcosa di totalmente nuovo e inaspettato, un nemico subdolo, un nemico invisibile, che ha sconvolto le nostre vite e che tutt'oggi ci lascia una contabilità di vittime che definire drammatica è dire poco. Ogni giorno leggiamo un bollettino che ci ferisce; molti di noi si sono ammalati, io stessa mi sono ammalata. Molti sono fortunatamente guariti, altri non ce l'hanno fatta; in questo momento, mentre noi stiamo discutendo dello scostamento di bilancio, ci sono i nostri meravigliosi operatori sanitari che lottano per salvare vite. In questo stesso momento, per le decisioni difficili che abbiamo preso in Italia, ma che sono state prese anche in altre parti del mondo e nel resto della stessa Europa, ci sono tanti che stanno soffrendo, che hanno incertezza e paura del loro futuro: i tanti che lavorano nel mondo delle imprese, i commercianti, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli artigiani, coloro che lavorano nel mondo dello sport, i tanti giovani che guardano a cosa accadrà nel loro futuro. Questo scostamento di bilancio che cos'è? È un'ulteriore prova di resistenza del nostro Paese, un'ulteriore prova della sua capacità di mettere in campo misure per sostenere chi oggi sta soffrendo. Sono previsti infatti nuovi interventi a tutela del lavoro e per il sostegno agli enti locali, alle Forze dell'ordine, al sistema di Protezione civile. Sono previsti stanziamenti aggiuntivi per il settore sanitario e per il sistema dei trasporti pubblici, al fine di garantire maggiore sicurezza e fronteggiare quindi la diffusione del virus. Sono previste le rimodulazioni temporali dell'invio delle cartelle esattoriali in favore delle imprese; misure che consentono di accelerare e potenziare la ripresa dell'attività economica. Si è tenuto conto della cosiddetta logica di filiera: il Governo ha aiutato tutte quelle attività che, seppur non formalmente chiuse, hanno subito cali di fatturato. Inoltre è stata data una risposta importante ad autonomi e partite IVA, sgravandoli di tutta una serie di oneri contributivi. Per rispondere a chi dice che questo Governo ha prodotto una quantità infinita di decreti volti a sistemare dimenticanze o orrori generati con tutti gli atti precedenti, mi corre l'obbligo di sottolineare che si tratta di dichiarazioni assolutamente false e tendenziose. i decreti emanati ed elaborati minuziosamente, accogliendo le osservazioni che via via le categorie e i cittadini ci hanno inviato, sono il frutto della continua e imprevista evoluzione di questa pandemia, che ci ha colpiti da un punto di vista sanitario e poi economico. È facile stare dall'altra parte, puntare il dito e giudicare. *(Applausi)*. È facile parlare senza rendersi conto che quella che stiamo vivendo è una situazione drammatica, senza soffermarsi sul fatto siamo stati messi di fronte a una condizione mai vissuta prima e per cui è stato necessario adottare misure che sono apparse drastiche, ma che in realtà erano semplicemente adeguate e proporzionate per tutelare il diritto alla vita, alla salute dei cittadini e a contenere la diffusione del contagio Il nostro Governo ha sempre agito sulla base delle valutazioni del comitato tecnico-scientifico scegliendo sempre la linea della trasparenza e della verità senza alimentare diffidenza e complottismo. Del resto, la verità è l'antidoto più forte; la trasparenza è il primo vaccino di cui dotarsi. *(Applausi)*. I primi tre scostamenti votati nel 2020 hanno messo in campo 100 miliardi. In occasione della legge di bilancio abbiamo votato un altro scostamento di altri 22 miliardi. Oggi, in vista del quinto decreto ristori, siamo chiamati a votare un ulteriore scostamento di 32 miliardi. Colleghi, parliamo di risorse fresche aggiuntive per oltre 150 miliardi rivelatesi fondamentali non solo per proteggere la nostra sanità, i nostri lavoratori, le nostre imprese, le nostre famiglie, ma anche per aprire convintamente una strada di sviluppo, per far trovare il Paese pronto a sfruttare tutte le potenzialità della ripresa del *recovery plan* una volta che ci saremo lasciati alle spalle questo complicato momento. Potevamo fare meglio e di più? Tutto si può e si deve migliorare, soprattutto in una fase storica così convulsa, ma colleghi non possiamo non avere l'onestà intellettuale di riconoscere la quantità e la qualità dello sforzo profuso. A tal proposito, vorrei fare giusto qualche esempio non con l'intento di esibire la lista della spesa, ma per ristabilire una necessaria verità rispetto a qualche narrazione disfattista e strumentale che pure in quest'Aula abbiamo dovuto ascoltare. dati Unioncamere di fine ottobre ci hanno detto che tra luglio e settembre 2020 il superbonus al 110 per cento, misura ideata e fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, ha fatto nascere più di 5.000 imprese edili. dati Unioncamere dei giorni scorsi certificano che nel 2020 il saldo generale tra imprese cessate e costituite è positivo: nonostante la crisi, ci sono 19.000 imprese in più, a dimostrazione dell'efficacia delle misure del Governo a supporto della resilienza del nostro tessuto produttivo. dati della Ragioneria generale e dell'Istituto sulla finanza locale dimostrano come gli investimenti nei Comuni proseguano a ritmo serrato: nei primi sei mesi del 2020 sono stati spesi 4 miliardi di euro in investimenti, il 17,4 per cento in più rispetto al 2018. «Il Sole 24 Ore» attribuisce tale merito alla cosiddetta dal MoVimento 5 Stelle, una norma che potrà produrre effetti ancora maggiori nei prossimi mesi. I dati Istat di due giorni fa certificano l'efficacia del patto per l'*export* messo in campo dal Ministro degli affari esteri: abbiamo il nostro *made in Italy* che dal novembre 2020 sale del 4 per cento in più al mese e dell'1 per cento in più rispetto a un anno fa. *(Applausi)*. I dati INPS riferiti alle ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ci dicono che a novembre 2020 sono state autorizzate oltre 173 milioni di ore e si riferiscono quasi interamente alla causale Covid-19. *(Applausi)*. A novembre del 2019 le ore autorizzate erano poco più di 14 milioni. Questo dato parla chiaro sugli sforzi effettuati dal Ministero del lavoro e dall'INPS. Non abbiamo abbassato lo sguardo - e lo dico in qualità di Presidente della Commissione lavoro sul contrasto alle discriminazioni di genere *(Applausi)*, sull'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani e delle persone con disabilità anche intellettive, sul riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. Sarà centrale migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, nonché delle micro-imprese italiane, in ritardo rispetto a quelle degli altri Paesi europei. Ridurre i divari tra i cittadini e i territori: questa è la vera opportunità per riprendere a investire, attivando potenziali di crescita e innovazione inespressi per creare opportunità di buon lavoro, in particolare per i giovani e le donne nei territori più marginali. Sviluppare un piano per le nuove competenze, prevedere attività di sostegno all'imprenditoria femminile, potenziare l'apprendistato duale e il servizio civile universale, investire in infrastrutture sociali, famiglia, comunità e terzo settore: questi sono i punti salienti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la parte «Inclusione e coesione». *(Applausi)*. Il grande senso di responsabilità e la solidarietà messe in campo dai nostri cittadini spingono anche noi, che abbiamo l'onore di servire il Paese, a fare tutto il possibile, mettendo a disposizione maturità, fermezza e capacità di visione perché, di fronte alla peggiore emergenza che l'Italia si è trovata ad affrontare da 70 anni a questa parte, è necessario dare supporto e sollievo ai nostri concittadini, tenendo ben saldo il timone dei valori costituzionali. Mi dispiace dirlo, ma qualcuno ha messo a rischio... I cittadini ci chiedono risposte e noi stiamo lavorando in questa direzione. Non c'è tempo da perdere, perché in questo momento i tempi della politica non coincidono con i tempi dell'emergenza, che necessita di velocità e di efficacia. Non dobbiamo perdere la connessione con la realtà, non dobbiamo farci distrarre da polemiche sterili. Fuori da quest'Aula ci sono milioni di persone che stringono i denti e che tengono duro, in attesa di tempi migliori. Per questo dobbiamo lavorare, affinché i ristori arrivino il prima possibile. Dobbiamo difendere a tutti i costi il nostro futuro, dando una prospettiva

Passiamo alla votazione.

parere favorevole del Governo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

di una lettera di un signore che si definisce un ex imprenditore del *fitness*, indirizzata al nostro Presidente della Repubblica e a tutti voi: «Buongiorno Egregi, sono qui a scrivervi la mia storia che poi è quella di molti altri. Dopo anni passati sui libri, nel 2006 ho iniziato la mia carriera imprenditoriale nel mondo delle palestre, piscine e sport in genere. Investimenti iniziali importanti, crisi economica del 2008, problematiche e difficoltà varie superate, attività a pieno regime per gli anni a seguito, fino a febbraio 2020. Dopo quattordici anni di fatica e di sudore, aperti tredici ore al giorno, vanto nessun debito tributario, nessuna tassa scavallata. Dal marzo 2020 al 31 dicembre 2020,

3.840 euro unici aiuti ricevuti per chiusure marzo, aprile e maggio. Solo terrore seminato e mai nessun incentivo per far ritornare le persone in palestra. Oltre 300.000 euro di perdite e mancati incassi che si ripercuoteranno per i prossimi quattro o cinque anni. Nessuna previsione certa di riapertura al 100 Ora, dopo tutto l'esborso di denaro per riuscire a rimanere in piedi fino ad oggi, io dovrei continuare a pagare gli affitti dei mesi di chiusura, le spese, le utenze, sperando di poter riaprire, forse, non si sa quando, dovendo poi far recuperare novembre, dicembre e gennaio con ingressi contingentati. Ma voi avete idea di quanto possa costare la gestione di un impianto sportivo e di una piscina? Vi ricordo che tutto questo non è causa di un'errata gestione imprenditoriale, ma è stato imposto e concordato dal Governo per tutelare e per salvare le vite di tutti gli italiani, comprese le vostre. Fosse almeno servito per sconfiggere il virus». Concludo con una frase che mi ha colpito: «Mio figlio Mattia di dieci anni mi chiede da mesi perché la palestra e la piscina di papà sono vuote. Io, ridendo, gli rispondo che sono tutti in coda dal tabaccaio a comprare le sigarette, eppure il fumo provoca circa 90.000 morti all'anno in Italia, ben più del Covid. Ora mi aspetto da voi politici almeno una risposta migliore della mia